La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche e integrazioni al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 29 marzo 2007. Anzitutto l'ordine del giorno di oggi pomeriggio è stato integrato con l'esame delle due ratifiche di accordi internazionali con la Francia e la Polonia, già previste dal calendario della settimana scorsa, che saranno esaminate a conclusione del dibattito sul programma legislativo europeo. La seduta potrà proseguire fino alle ore 20,30. Nella giornata di domani sarà discusso il decreto-legge in materia di attuazione di obblighi comunitari e internazionali che, ove non concluso, potrà eventualmente proseguire nel pomeriggio di martedì 20 marzo. È stato infatti confermato di dedicare l'intera seduta antimeridiana di giovedì 15 marzo alle mozioni sulla politica ambientale. A inizio della seduta antimeridiana di mercoledì 21 marzo si procederà ad una unica chiama dei senatori per la elezione, mediante schede, di due senatori Segretari ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del Regolamento, e di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 12,30. Nella stessa giornata di mercoledì 21 inizierà l'esame del decreto-legge recante proroga di missioni internazionali, ove concluso dalle Commissioni riunite 3a e 4a. L'eventuale seguito della discussione generale potrà avvenire nella seduta antimeridiana di martedì 27 marzo, da convocare se necessario a tal fine. Le votazioni avranno inizio - auspicabilmente per concludersi - nella seduta pomeridiana di martedì 27 marzo. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

marzo, nella mattinata, si terrà in Aula la manifestazione ufficiale, alla presenza delle delegazioni dei vari Parlamenti europei. Il calendario della prossima settimana - fin da martedì 20 marzo, se l'*iter* del decreto-legge sugli obblighi comunitari lo consente - prevede inoltre la discussione di tre mozioni: sull'accattonaggio minorile, sugli ufficiali di Marina in ferma prefissata e sull'industria conserviera del pomodoro, con eventuale prosieguo nella settimana successiva. Tra il 28 e il 29 marzo, saranno inoltre posti all'ordine del giorno il decreto-legge in scadenza in materia di liberalizzazioni, tuttora all'esame della Camera dei deputati, e ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente.

*relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'integrazione ha il significato di sviluppare e sottolineare alcuni aspetti importanti sia di procedura che di Volevo appunto segnalare come noi sviluppiamo la nostra discussione sull'esame del programma legislativo di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e del programma di 18 mesi delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena, tra il Consiglio europeo dell'8‑9 marzo e il 25 marzo, quando sarà celebrato a Berlino il 50° anniversario dei Trattati di Roma. Nel Consiglio dell'8-9 marzo è stata rilanciata la Strategia di Lisbona e nel vertice susseguito si è raggiunto un importante accordo sulle questioni ambientali e climatiche per ridurre i gas serra e sviluppare le energie rinnovabili. Questo è un segno di grande vitalità dell'Europa, che può mettere il nostro continente all'avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici, grazie alla coesione degli Stati. Il 25 marzo, cioè tra pochi giorni (come ha detto il presidente Marini, il 23 marzo ci sarà una celebrazione presso la nostra la nostra istituzione), sarà adottata un'importante Dichiarazione per il futuro dell'Unione Europea, su cui sta lavorando il cancelliere tedesco, nonché presidente di turno, Angela Merkel, che, a quanto si sa, verterà su alcuni punti fondamentali, cioè sui successi del passato dell'Unione Europea, sui valori comuni europei e sugli obiettivi per il futuro, in primo luogo i problemi dello sviluppo, della difesa, dell'energia e i grandi impegni relativi alle questioni istituzionali. Il 21 e 22 giugno 2007 si terrà il Consiglio europeo in cui si discuterà degli sviluppi futuri del Trattato costituzionale. Ho voluto citare queste date per sottolineare il lavoro serrato che si sta svolgendo a livello europeo e ricordare a tutti noi il momento ancora

da parte di tutti noi, l'esigenza di un rilancio dell'Europa. Tutti avvertiamo la necessità e l'importanza di un rilancio dell'unità europea e, al contempo, l'esigenza di dare ad essa un'anima, di farla avvicinare alla gente. Ecco, questo è stato un po' - lo volevo

di una risoluzione di carattere procedurale, nel senso che rappresenta una cornice unitaria in cui sviluppare il nostro confronto, pur conoscendo le diversità di opinioni che ci sono tra noi e che sono note.

divisioni su punti contingenti, magari già discussi nella scorsa legislatura e collegati solo alla nostra polemica interna, dobbiamo offrire all'Europa la comune volontà del Parlamento italiano di favorire gli sforzi che si stanno facendo per garantire all'Unione Europea un futuro certo e importante.

l'India il 12 per cento, gli USA scenderanno dall'attuale 29 al 15 per cento. In questa prospettiva, i Paesi europei possono svolgere un ruolo da protagonista solo se esiste un'Europa forte e coesa. Queste considerazioni rafforzano il senso politico della nostra discussione in Commissione, la quale si è soffermata sui punti più qualificanti che derivavano dai due documenti programmatici in esame; tra questi, assume importanza rilevante il tema della riforma istituzionale. In questo senso si è ritenuto di indirizzare l'azione del Governo con questa risoluzione, in vista del prossimo 25 marzo e del prossimo Consiglio di giugno, fondamentalmente con una con una indicazione importante, per fare tutto ciò che è possibile al fine di concludere positivamente il processo costituzionale europeo. Su questo tema, come sapete, in questi giorni, subito dopo la stessa Commissione, vi sono stati importanti interventi. Angela Merkel ha ricordato,

l'Europa è caratterizzata dalla sua molteplicità e dalla sua diversità: un patrimonio che deve essere tutelato dalla libertà (io

getti le basi per nuove regole comuni che permettano all'Europa di affrontare queste sfide, quindi di essere operativa e di essere ampliata. ha annunciato un piano di consultazione dei Capi di Stato e di Governo al fine di cercare di trovare una soluzione che consenta di uscire dalla stasi odierna e, successivamente, proporre al vertice di giugno una tabella di marcia per il varo del nuovo trattato. Tali consultazioni dovranno portare a nuove regole prima delle prossime elezioni europee. Penso che questo sia molto importante. Per quanto ci riguarda, vorrei ricordare l'intervento del ministro D'Alema, secondo cui un accordo è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per rilanciare l'Europa.

innovazioni introdotte nel Trattato costituzionale (un Ministro degli esteri che presieda la Commissione affari generali del Consiglio e faccia parte della Commissione, un Presidente stabile del Consiglio europeo, l'estensione del voto a maggioranza qualificata, l'adozione della Carta europea dei diritti fondamentali). Tuttavia, egli dice, l'accordo dovrà anche prevedere una decisione esplicita sui confini esterni dell'UE, nonché una revisione molto più rapida delle politiche dell'Unione e delle risorse finanziarie, che devono essere all'altezza dei problemi globali. Una posizione condivisa fondamentalmente, in diversi modi, anche da altri esponenti europei. In questo senso ci pare importante ribadire quello che abbiamo detto, cioè trovare il modo affinché entro il 2009 si possa risolvere il problema importante del Trattato costituzionale. Per quanto riguarda il resto, e mi avvio a conclusione, i due programmi mirano a rispondere alle attese dei cittadini e a far fronte alle sfide comuni con le quali l'Europa si deve confrontare, tra le quali, come detto e ripetuto continuamente, la globalizzazione, il cambiamento climatico, il problema energetico, il terrorismo nazionale, la questione della guerra e della pace. Per la prima volta, la Commissione ha definito una serie di azioni concrete, le cosiddette iniziative strategiche, che rappresentano il fulcro del suo lavoro per il 2007. Queste iniziative vertono su quattro obiettivi che riprendo per comodità di discorso: rimettere l'Europa sulla via della prosperità economica (è un punto importante nel momento in cui c'è un nuovo ciclo di sviluppo economico che vede l'Europa crescere positivamente, compreso il nostro Paese), rafforzare l'impegno a favore della solidarietà e della coesione sociale, migliorare la sicurezza dei cittadini, rafforzare la dimensione mondiale dell'Europa. Scorrendo la relazione, si vedranno, e rinvio ad esse, le proposte specifiche sul versante della modernizzazione dell'economia europea secondo le linee fondamentali che mirano a favorire la crescita sostenibile e l'occupazione nel quadro della nuova fase della Strategia di Lisbona. Inoltre, enumero l'iniziativa a favore delle imprese, della piccola e media impresa, della ricerca, ma anche le iniziative, la preoccupazione tesa a rispondere alla domanda di sicurezza e di coesione sociale, molto sentita in tutti i Paesi. Su questo punto c'è stata anche tra noi una discussione importante e ritengo questo questo uno dei punti cardine su cui si deve costruire l'Europa dei diritti, che deve coniugare libertà e sicurezza. D'altronde, questo è un tema di fondo che ci hanno consegnato i *referendum* francese e olandese, a cui occorre rispondere senza nascondere i problemi. Un altro punto importante che vorrei sottolineare (mi sembra si stia discutendo in questi giorni non solo nell'agenda, ma nello sviluppo stesso dell'iniziativa, in primo luogo, del Presidente tedesco) è l'approvazione del Piano di azione europea in materia di politica energetica. La Presidenza tedesca si è impegnata alla completa apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, prevista per il 1° luglio 2007, garantendo un'implementazione unitaria di tutti gli Stati membri delle direttive comunitarie. È molto importante che sia andata avanti l'iniziativa della lotta contro l'inquinamento e il cambiamento climatico; essa, in effetti, è diventata una delle priorità della Presidenza. Penso che proprio attorno a ciò, con la decisione di abbassare del 20 per cento i gas serra, noi ci poniamo, e lo voglio ribadire come all'inizio, in termini molto forti e precisi, in una logica di grande guida del processo politico e dello sviluppo del Paese. Per quanto riguarda le questioni internazionali, mi sembra che, secondo le linee guida contenute nella Strategia europea di sicurezza, adottata il 12 dicembre del 2003 dal Consiglio europeo, nei Paesi confinanti con l'Europa l'impegno delle tre Presidenze sarà principalmente volto alla stabilizzazione dei Balcani occidentali. Lo ripeto perché oggi mi sembra che, dopo il dopo il fallimento della trattativa sul Kosovo, ci sia bisogno di maggiore attenzione e la questione dei Balcani occidentali, per quanto ci riguarda, deve diventare prioritaria insieme ad altre, ma certamente con un'attenzione in più rispetto allo stato rispetto allo stato di principio che è stato esposto nei programmi delle tre Presidenze. Saranno anche rafforzate in questo senso

Sarà inoltre considerato prioritario il rafforzamento del partenariato con la Russia nell'ambito dei quattro «spazi comuni» e l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione. Le future Presidenze si impegnano a mantenere il sostegno dell'UE a favore della pace e della stabilità, in particolare attraverso la cooperazione con l'ONU e con la NATO. Sarà posto l'accento sull'assistenza nei settori della prevenzione dei conflitti, della ricostruzione e stabilizzazione postconflitti e della giustizia di transizione. La Presidenza tedesca sarà a favore di un'ulteriore stabilizzazione della situazione in Libano. Quindi, c'è la decisione di seguire positivamente l'iniziativa già avviata con UNIFIL in Libano, di cui il nostro Paese è stato anche portatore; dunque, l'Europa mantiene e sostanzia

un aiuto al rilancio del progetto europeo, all'esigenza di un'Europa come luogo in cui il nostro Paese, il nostro Continente, possa agire positivamente

a partire anche dalle nostre diverse posizioni, dare un contributo forte al dibattito, al prossimo 25 giugno, al prossimo Consiglio europeo, perché l'Italia lo può fare: è uno dei Paesi che maggiormente ha voluto l'Europa e dobbiamo continuare a farlo.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, cinquant'anni or sono si consolidava, con i Trattati di Roma, il progetto politico della Comunità economica europea, forse una risposta debole a fronte di più incisive soluzioni ipotizzate, ma un progetto rivoluzionario negli scopi e ben ponderato nei metodi. Un progetto di pace e di sviluppo, di pace attraverso lo sviluppo e di sviluppo attraverso la pace. Rispetto delle differenze, partecipazione, condivisione delle scelte, sussidiarietà, solidarietà sono i principi che hanno decretato il successo del nostro Continente e quello del nostro Paese, che nell'Europa ha creduto e che con l'Europa è cresciuto in benessere e democrazia. L'Europa è la dimostrazione di quanto si possa realizzare con il dialogo, con la reciproca conoscenza, valorizzando ciò che ci unisce all'altro più di ciò che ci separa da lui: è una rivoluzione profonda che ha trasformato concetti giuridici e assiomi politici che sembravano intoccabili ed eterni: la sovranità, i confini, la moneta. È un processo che ha inciso e incide sulla nostre coscienze di cittadini, di persone, puntando al nostro orizzonte di vita, il nostro spazio sociale, la nostra cultura. Oggi l'Europa è una realtà che coinvolge 27 Paesi e alla quale altri popoli aspirano ad unirsi. Purtroppo l'arresto del processo costituente ci fa oggi vivere una nuova *impasse*. L'entrata in vigore del Trattato costituzionale è un'esigenza primaria, è essenziale un nuovo slancio istituzionale dell'Unione Europea, una sua implementata visione in un momento storico in cui l'Europa è cresciuta, ha bisogno di visibilità e credibilità sulla scena mondiale. È urgente, e l'apertura di nuove negoziazioni sarebbe antistorica e pericolosa. Peraltro, se da un lato dobbiamo impegnarci per il successo del Trattato, dall'altro non dobbiamo ignorare le ragioni che hanno permesso di rallentare la costruzione europea. Sono ragioni che risiedono negli scarsi sforzi fatti finora per associare i cittadini alle scelte dell'Europa; un'Europa in cui ci sono ancora troppo Stato, troppa burocrazia e troppo poca democrazia diffusa; un'Europa che decide lontano dai cittadini, attuando scelte talvolta incomprese perché non condivise né partecipate. Il ruolo degli Stati e dei Parlamenti nazionali nella soluzione del*deficit* democratico europeo è dunque basilare nel quadro di un nuovo processo che stimoli le coscienze dei cittadini europei e riconosca loro e alle articolazioni *sub*-statali nelle quali sono organizzate il necessario ed adeguato peso decisionale. È vitale perché l'Europa riparta con nuovo vigore, restando fedele ai suoi principi originari di rispetto e valorizzazione delle differenze di quelle tante tessere che compongono questo magnifico mosaico; è necessario perché le azioni programmate dalla Commissione e dalle Presidenze europee non incontrino ulteriori ostacoli ed anzi si completino grazie all'apporto fattivo dei cittadini, dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Sicurezza, ambiente, energia e sviluppo economico sono le grandi sfide che ci attendono. Come possiamo pensare di confrontarci con queste sfide globali se prima non perfezioniamo la nostra architettura istituzionale, se prima l'Europa non si rafforza al suo interno? Malgrado le difficoltà, l'Europa non si è persa d'animo; lavora per produrre realizzazioni concrete in favore dei suoi cittadini, per cancellare quel velo di ermetismo burocratico che ancora troppo caratterizza le sue norme e i suoi procedimenti. Il programma della Commissione per il 2007 lo testimonia con le priorità stabilite per modernizzare l'economia europea, per completare il mercato interno, per l'approvvigionamento ed una corretta gestione delle risorse energetiche, per una migliore gestione dei flussi migratori con quelle in favore della ricerca, in materia di sicurezza e di giustizia, di cooperazione e di relazioni di vicinato, di reti e di trasporto. Sono punti qualificanti, ma forse ancora più importanti, perché mirano a promuovere un'Europa delle coscienze, lo sono gli interventi in materia di lavoro e occupazione, di strategia sanitaria, di istruzione e cultura, di politiche sociali, di comunicazione e trasparenza, di semplificazione normativa e di sburocratizzazione. La Commissione ha ben compreso: se le sfide istituzionali e costituzionali non possono essere ignorate, è altrettanto vero che esse possono essere affrontate solo attuando in parallelo un programma politico che si concentri sulle attese e sulle esigenze dei cittadini. I risultati concreti faranno aumentare la fiducia nel progetto europeo e creeranno le condizioni favorevoli per addivenire ad un accordo istituzionale ambizioso: avvicinare l'Europa ai cittadini, permettere ai cittadini e alle articolazioni *sub*-statali di agire in Europa e per l'Europa affinché l'Europa mantenga e rafforzi la sua vitalità. Questa, dunque, è la nostra priorità. Credo che tutto possa riassumersi nella realizzazione di pochi principi. Il primo riguarda innanzitutto trattare situazioni diverse secondo regole adeguate e diverse, non è mettere in discussione l'unità; anzi, allontanando i rischi di imposizione, si consolidano proprio quella omogeneità e quella coesione interna necessaria all'Europa. alla montagna; non è possibile continuare ad ignorare le sue specificità credendo di poter estendere alla montagna le stesse regole valide per le aree urbane o per le pianure. Le sue peculiarità climatiche, orografiche e culturali richiedono un'attenzione particolare, richiedono costi sostenuti in servizi perché questi territori possano essere mantenuti, possano continuare a garantirci dai rischi ambientali; richiedono interventi per poter attrarre attività in grado di assicurare uno sviluppo durevole, in grado di creare occupazione e benessere. La montagna non è semplicemente un luogo di divertimento e vacanza; non è una zona di passaggio (penso alle valli alpine e alla mia Regione, la Valle d'Aosta) dei flussi commerciali su gomma. È uno spazio vissuto e che deve poter continuare a vivere in prosperità. Banalizzare la montagna, non assicurarle risorse e strumenti normativi adeguati, impedire o non favorire la piena esplicazione dell'autonomia istituzionale e finanziaria delle Regioni e degli enti locali cui compete la responsabilità di governo di questi territori è un grave errore, con possibili conseguenze negative per l'Italia e per tutto il continente. Il Governo e il Parlamento devono riconoscere appieno queste peculiarità e continuare nella loro attività di sensibilizzazione a livello europeo, allo scopo di riconoscere alla montagna il giusto ruolo, la giusta posizione in Europa e la dovuta autonomia. Anche le diversità culturali, istituzionali, costituzionali e storiche sono da considerare. Le Regioni e le Province autonome sono confrontate alle scelte e alle decisioni prese a livello europeo, spesso in contrasto con le loro aspettative e con le loro prerogative; il tutto senza aver potuto validamente partecipare a queste scelte e a queste decisioni. È evidente che in tale situazione l'Europa è percepita come lontana, quando non come un avversario. Voglio citare una recente esperienza della mia Regione, la Valle d'Aosta, che si è vista imporre la cancellazione dei benefici derivanti dall'esenzione fiscale su alcuni contingenti di beni: è un segnale di queste disfunzioni. È difficile per noi comprendere una decisione che ignora le prerogative costituzionali della Regione, perché di questo si è trattato. Un diritto storico, riconosciuto ai valdostani e sancito costituzionalmente, viene annullato d'incanto, senza che la Valle d'Aosta abbia avuto voce in capitolo e senza che questo diritto, vigente, avesse comportato conseguenze percepibili sul funzionamento del mercato interno. Sto parlando di una Regione che, per la sua cultura bilingue, la sua posizione frontaliera e la sua millenaria tradizione di autogoverno, ha sempre guardato all'Europa in termini assolutamente positivi e che alla costruzione europea ha fattivamente partecipato, anche attraverso numerose iniziative di cooperazione transfrontaliera ed interregionale. Non credo che simili decisioni rafforzino l'Europa delle coscienze. È necessaria una maggiore attenzione a queste situazioni. È necessario un potenziamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome e della loro partecipazione alle decisioni europee, in tutte le materie di loro competenza, per tutte quelle materie ed iniziative (penso all'ambiente e ai trasporti) che possono impattare sul loro quotidiano e sul loro sviluppo. Urge, in tal senso, un deciso e forte intervento del Governo e del Parlamento, per ragioni di democrazia e di diritto, in favore dell'Europa. Partecipazione alle scelte, dunque, come secondo principio, che non può prescindere dall'essere presente al Parlamento europeo. Ogni Regione, ogni Regione a Statuto speciale ed ogni Provincia autonoma deve avere almeno un proprio rappresentante in quella sede, per apportarvi il proprio contributo di realtà peculiare, per comprendere le esigenze dell'Europa e per rappresentare le proprie esigenze d'Europa. Anche in quest'ambito, urge un deciso e forte intervento del Governo e del Parlamento. In conclusione, il nuovo slancio di cui necessita il progetto europeo passa necessariamente attraverso il consolidamento interno dell'Unione, che deve operare per sviluppare la conoscenza e la coscienza dell'Europa nei cittadini e nella società. Non possiamo ignorare questa esigenza e questo messaggio. Come Parlamento e come Governo dobbiamo consacrare ogni possibile sforzo affinché l'Europa non sia il pretesto per imporre scelte mortificanti per la nostra comunità e le nostre autonomie. Dobbiamo vegliare e operare affinché l'ambizioso obiettivo sia realizzato: quello di un'Europa che sia il grande spazio democratico di canalizzazione positiva delle diversità, di benessere e di sviluppo voluto dai Padri fondatori. Queste credo siano le garanzie che dobbiamo dare ai nostri cittadini, alle nostre Regioni, questo è il patrimonio che l'Italia deve portare in dote al prossimo Vertice di Berlino.

Ho particolarmente apprezzato l'impegno richiesto dal relatore affinché il Senato e il Parlamento italiano portino un aiuto alla ripresa del progetto europeo. La costruzione europea si avvicina al suo ennesimo appuntamento con la storia; il *focus* è centrato sulla Presidenza tedesca in vista del del vertice del 25 marzo a Berlino nel Cinquantenario dei Trattati di Roma. Girata, poi, la boa delle elezioni francesi, il Consiglio del 21 e 22 giugno dovrà tracciare la *road map* per la riattivazione del processo costituente, con la previsione che i risultati programmati dalle tre Presidenze si colgano dopo di esse - nel secondo semestre 2008, appunto - con un altro giro di boa sotto la Presidenza francese. Dunque, siamo alle mosse di partenza di un percorso decisivo. Il cancelliere Angela Merkel ha ottenuto, a quanto si è letto, il consenso di massima dei suoi 26 colleghi allo schema della Dichiarazione di Berlino, che prevede cinque paragrafi sulla cooperazione europea vista nell'arco del cinquantennio (risultati, caratteri, valori, priorità, impegni) senza, al momento, chiamare direttamente in causa il Trattato costituzionale che alcuni vorrebbero ribattezzare come «istituzionale» o «fondamentale». A quanto se ne capisce - ma, certo, il ministro Bonino può darci ragguagli assai migliori di quelli di cui io potrei essere capace - a Berlino si intende anzitutto confermare solennemente i risultati storici conseguiti, i connotati istituzionali raggiunti, i valori di riferimento; poi, sulla base di quelle acquisizioni da ritenersi ormai da tutti irrinunciabili, definire una scala di priorità e di impegni di cui al momento è chiara soltanto la scadenza che deve precedere o coincidere con le elezioni europee del 2009. quale deve essere in proposito l'indirizzo del Senato della Repubblica? Il Governo ha individuato nella costruzione europea il punto prioritario delle proprie relazioni internazionali e delle sue stesse politiche interne su scelte di grande portata: la dimensione europea nella cooperazione strategica per la sicurezza e la pace, nella diversificazione energetica e nella protezione ambientale, la dimensione europea nelle infrastrutture di comunicazione (materiali e immateriali), ed anche gli obiettivi economici e sociali dell'Agenda di Lisbona, la collaborazione in materia di giustizia e di sicurezza interna, le politiche di liberalizzazione (aperture dei mercati, tutela della libertà di concorrenza). Qual è la svolta del cinquantennale? Credo sia una svolta dettata dall'evidenza che si coglie ogni qual volta l'Europa guarda non dentro di sé, ma fuori di sé; l'evidenza del quadro globale indica che l'Unione Europea, Europea, che 50 anni fa era un'azzardata scommessa, oggi è uno stato di necessità. Si tratti della costruzione della pace nel Medio Oriente, della competizione con i capitalismi asiatici o dell'azione universale per i diritti umani, l'Italia - come ogni altro Stato dell'Unione - è di per sé uno Stato minore perché il formato degli Stati nazionali non può corrispondere alle dimensioni dei problemi globali. Se la costruzione europea non è più una scommessa ma una necessità, si impone allora di porre termine alla pausa di riflessione che è seguita - e dura anche troppo - agli insuccessi dei *referendum* francese ed olandese; si impone di riattivare il cammino verso la cittadinanza comune. D'altra parte, il riconoscimento costituzionale dei diritti di cittadinanza comune è la condizione - ma forse avrebbe dovuto esserne il presupposto - perché si consolidi l'allargamento dell'Unione

ma entro il 2009 le due scale di grandezza si devono riequilibrare e devono essere compensate. Signor Presidente, muovendo da siffatte motivazioni, abbiamo promosso la costituzione, in entrambe le Camere,

per impegnare il Governo a contribuire alla Dichiarazione di Berlino senza accettare soluzioni minimaliste né compromessi al ribasso. Per esigenze di Regolamento (essendo ormai, con la discussione di oggi, alle soglie dell'appuntamento di Berlino), abbiamo trasformato quella mozione in un ordine del giorno che confidiamo il Governo vorrà accogliere per quanto lo concerne. Dico così perché l'ordine del giorno G1 non chiama in causa soltanto l'azione di Governo, ma si rivolge anche alla pubblica opinione rivendicando alla cittadinanza europea la possibilità di esprimersi direttamente circa il riconoscimento costituzionale dei propri diritti. È in via di attuazione in tutta l'Unione Europea la sottoscrizione di un milione di firme sotto la petizione che chiede il *referendum* consultivo in contemporanea con le elezioni europee del 2009, affinché il Trattato costituzionale riceva il consenso unitario e diretto del *demo**s* europeo che, se fosse così consultato, potrebbe provvedere direttamente a ripianare il proverbiale *deficit* democratico dell'Unione ed anche ad autocertificare la propria contestata esistenza. In relazione al comunicato del ministro D'Alema rilasciato se davvero una rapida conferenza intergovernativa arrivasse alla ratifica definitiva del Trattato prima delle elezioni europee del 2009, non sarei per niente dispiaciuto che l'iniziativa del *referendum* fosse oltrepassata dai fatti. In attesa che ciò accada, crediamo utile sostenere l'idea del *referendum* come sentenza di appello affidata al giudice naturale. Ladifficoltà dell'impresa non ci sfugge, ma riteniamo che il sostegno al *referendum* richiesto dai federalisti sia anche, da parte del Senato, il modo di rendere onore al centenario della nascita di Altiero Spinelli e al cinquantenario del suo Manifesto dei Federalisti europei (recentemente ristampato nell'edizione anastatica del 1957). In quel manifesto, significativo per la sua datazione in quanto contemporaneo ai Trattati di Roma, Spinelli non si mostrava tenero, com'è noto, verso i Governi nazionali e neanche verso i partiti degli Stati nazionali, ai quali rimproverava - citazione - «il rifiuto sistematico di prendere in considerazione anche solo l'ipotesi di dare la parola al popolo europeo». Oggi si è data qui l'occasione di riscattarsi dal rimprovero di Spinelli e di prendere quell'ipotesi in considerazione. L'ordine del giorno che presentiamo al Senato questo chiede: che il popolo europeo possa essere chiamato a decidere sulle proprie istituzioni comuni, sui propri diritti individuali, sulla propria cittadinanza, non ricevuta per retaggio ma liberamente voluta come patto costituzionale. Se non ci si arriva prima del 2009, deve essere il popolo europeo a decidere.

ha subito un incidente molto spiacevole, direi serio, ma le ultime notizie sono rassicuranti. La Commissione che presiedo, e della quale egli fa parte, gli ha formulato un sincero augurio di pronta guarigione. Ritengo opportuno opportuno che anche l'Assemblea sia informata e gli rivolga coralmente un augurio. Abbiamo bisogno che il collega Mantovano torni presto in quest'Aula perché abbiamo bisogno del suo lavoro così serio e così apprezzato. *(Applausi)*. ringrazio il collega Bianco e ne approfitto per dare informazioni di pochi minuti fa. Il collega Mantovano sta molto bene,

la situazione era tragica; per fortuna, con il passare delle ore, è diventata sempre meno tale e ho sentito direttamente Mantovano al telefono che mi ha detto che stava bene e che nella giornata di domani, al più tardi giovedì mattina, sarebbe stato addirittura dimesso dall'ospedale. Ringrazio

l'evoluzione delle sue condizioni fisiche; formuliamo a lui e alla sua famiglia tutti i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. Ripeto, le indicazioni che abbiamo parlano di una situazione in evoluzione: sono in corso accertamenti, quindi formulo a lui un augurio di pronta guarigione. finestra"). Sono certo di interpretare i sentimenti dell'Assemblea nell'inviare, a nome di tutti noi, un augurio di pronta guarigione sia al senatore Mantovano sia al senatore Micheloni.

se chiedessimo qual è l'immagine che c'è sull'euro probabilmente nessuno di noi se la ricorderebbe. C'era un tempo in cui la moneta rappresentava il volto dell'imperatore; in qualche modo era un volto dell'Europa. Ci siamo interrogati prima e in questi anni su quale sia il volto che vogliamo dare all'Europa.

parlando con una sola voce e riconoscendosi in grandi valori condivisi, che riflettono il ruolo storico e la sempre viva lezione ideale del Cristianesimo».

Veniamo da una comune eredità umana e cristiana» affermava il Presidente della Repubblica; in base a tale eredità dobbiamo «rivendicare una cultura ed uno spirito genuinamente europeo» per evitare che il patrimonio spirituale dell'Europa del XXI secolo si riduca a un sito archeologico. Giuliano Amato, allora vice presidente della Convenzione europea, pubblicamente riconosceva il valore identitario per l'Europa della religione cristiana e l'opportunità della sua inclusione come principio fondante nel testo della nascente Costituzione, alla cui natura aveva direttamente contribuito insieme al presidente Fini.

quale, come afferma Giovanni Paolo II «non riguarda solo gli uomini di scienza, così come non deve rinchiudersi nei musei». Anzi, essa «è la dimora abituale dell'uomo, ciò che caratterizza tutto il suo comportamento e il suo modo di vivere, persino di abitare e di vestirsi, ciò ch'egli trova bello, il suo modo di concepire la vita e la morte, l'amore, la famiglia e l'impegno, la natura, la sua stessa esistenza e la vita associata degli uomini». A questo principio e a queste radici comuni cristiano-giudaiche dobbiamo molto della nostra cultura laica, laica, del principio di separazione fra Stato e Chiesa e nel campo dell'arte con l'Europa delle basiliche e delle cattedrali; ad esse dobbiamo molto del principio del rispetto della dignità e della libertà umana umana e, Presidente, del rispetto della dignità di tutti gli uomini. Il principio di uguaglianza tra tutti gli uomini è un principio che nasce comunemente con la cultura cristiana e l'Europa sopravvive e l'Europa sopravvive all'Impero romano sulle strade stesse di quella che era Roma, portando questo nuovo fattore di unità. In un momento di disgregazione, in qualche modo la religione cristiana costituisce un collante e un continuo della storia romana e quindi un continuo di una storia di civiltà.

geografica e continentale potessero sommarsi degli altri elementi di Europa presenti nelle altre culture. Sono i concetti di Magna Europa di Henri Brugmans ed anche di un processo

«L'avventura, il dramma dell'epoca moderna, fu di aver conquistato il mondo dopo aver distrutto nella stessa Europa il principio di unità che avrebbe adesso permesso di organizzare la sua conquista. Un'Europa unita attorno al principio cristiano avrebbe potuto fare opera civilizzatrice: un'Europa un'Europa divisa in nazioni poteva fare solo opera colonizzatrice. Proiettando nelle altre parti del globo le sue divisioni religiose, i suoi conflitti politici, le sue rivalità economiche e, infine, le sue idee rivoluzionarie, l'epoca dell'uomo ha fallito il suo destino». Che errore di prospettiva, quando si dimentica di far entrare nelle storie dell'elemento coloniale la storia della stessa Europa! Signor Presidente, questo ordine del giorno

fra uomo e donna, di attuare non la divisione in censo ma il principio di uguaglianza di fronte alla legge e, prima ancora, di fronte a Dio.

Signor Presidente, onorevole Ministro, una ridotta attività parlamentare - come emerso anche in Conferenza dei Capigruppo - ha avuto tuttavia il pregio di ritagliare uno spazio per affrontare in Aula questioni rilevanti di politiche dell'Unione, valorizzando il ruolo del Parlamento rispetto ad importanti scadenze; tutto ciò in linea con gli obiettivi della legge La Pergola prima e Buttiglione poi, che hanno provveduto ad incrementare gli spazi a disposizione del Parlamento, prendendo coscienza dell'interdipendenza crescente tra ordinamento comunitario e nazionale. L'occasione è determinata dall'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2007 e sul programma di 18 mesi delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena. Ciò avviene immediatamente dopo la conclusione del Consiglio europeo di Bruxelles e a ridosso della cerimonia celebrativa di Berlino del 25 marzo per il cinquantenario della firma dei Trattati di Roma. Registriamo con soddisfazione il fiorire di iniziative che sia nel nostro Paese che in tutta Europa ricordano lo storico avvenimento. Nella risoluzione della Commissione Politiche dell'Unione è stata recepita l'indicazione del senatore Buttiglione di sviluppare una campagna di sensibilizzazione sulle ragioni e i valori dell'Europa in tutto il Paese, in particolar modo nelle scuole e nelle università. Di questo devo ringraziare il presidente Manzella, molto sensibile a questi temi. Riteniamo importante sottolineare questo aspetto al fine di far crescere nei giovani un forte sentimento europeo. Dobbiamo muovere oggi però dalle sollecitazioni del Presidente della Repubblica che, fin dal discorso del suo insediamento, ricordò che «l'Europa è per noi italiani una seconda Patria» e la necessità di superare la crisi che ha investito l'Unione dopo l'esito sfavorevole del *referendum* in due Paesi fondatori, come Francia e Olanda. Va superato allora il trauma di quel pericoloso deragliamento, riprendendo un cammino di integrazione tra popoli, economie e culture. Come possiamo non ricordare le considerazioni dello stesso presidente Napolitano nel recente intervento a Strasburgo, il 14 febbraio scorso, di lavorare per uscire dall'*impasse*, non dovendo ripartire da zero, dopo che 18 dei 27 Stati membri hanno già ratificato il Trattato in rappresentanza di 275 milioni di cittadini. Proprio la Francia di Giscard, presidente della Convenzione europea, ha preferito scadute illusioni ad un moderno realismo. L'Europa è oggi una moneta, è mercato, è insieme di istituzioni, è democrazia, è libertà, è diritti, è pace. Ma un'Europa di 27 popoli e 475 milioni di abitanti non può vivere senza Costituzione. È necessario allora riprendere quel percorso interrotto al fine di dotare l'Unione di istituzioni più forti, di nuove regole comuni per affrontare nuove sfide, con una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali, maggiore trasparenza nelle decisioni; per essere più operativa e funzionale nella sua nuova dimensione di Europa riunita. Non vi è dubbio che la prima questione che abbiamo di fronte è quella di impegnare il Governo a svolgere ogni azione per concludere positivamente il processo costituzionale europeo, riaffermandone i valori che sono alla sua base. Tutto ciò sarebbe importante che fosse realizzato prima della scadenza elettorale del 2009. Ancora una volta le elezioni europee potranno tenere sveglie le coscienze dei nostri popoli, obbligando l'Europa ad agire, come ripeteva Monnet. Particolare apprezzamento deve essere riconosciuto all'azione svolta dal cancelliere Angela Merkel, per il suo riconosciuto entusiasmo giovanile nel ritrovare l'anima dell'Europa. Non vi è dubbio che, rispetto alla validità dei programmi delle tre Presidenze che si succederanno nei prossimi dodici mesi, la necessità di riformare il Trattato è prioritaria, e dobbiamo fare ogni sforzo per evitare un fallimento che diventerebbe un errore storico. Bene ha fatto Angela Merkel a richiamare il modello sociale europeo, costruito in passato in una struttura demografica favorevole, che potrà essere difeso e salvaguardato nella sua generosità, senza mettere a rischio le conquiste sociali, solo se l'Europa saprà essere più competitiva e in grado di affrontare le sfide nuove della globalizzazione. Occorre tenere conto delle tendenze in atto in fatto di demografia, di tecnologia e di globalizzazione. Dal peso del 28 per cento sulla popolazione mondiale alla vigilia della Grande guerra si è progressivamente scesi al 13 per cento, perdendo centralità anche economica, che è diminuita dal 47 al 10 siamo a un livello inferiore al tasso di rimpiazzo. I figli vengono visti come una minaccia per il presente e non una speranza per il futuro. Non può essere dimenticato il grave problema del cambiamento demografico in Europa e le sue conseguenze in termini di natura economica e sulla società. Di qui la necessità di individuare risposte positive per le politiche verso la natalità, la maggiore dotazione di infrastrutturazioni sociali, l'intensificazione degli scambi e delle esperienze sulle politiche familiari. Particolarmente importante è l'impegno delle tre Presidenze, in specie quella tedesca, di creare «un'alleanza per le famiglie» nell'Unione, costruendo una solida piattaforma nell'azione di rafforzamento della famiglia, sui servizi di assistenza e cura dei bambini, anziani e disabili, conciliando i tempi della vita lavorativa e familiare, e l'impegno per un approccio integrato volto a garantire un ambiente favorevole alla famiglia. Sono indicazioni importanti che emergono. Le politiche familiari sono però essenzialmente di competenza nazionale. A tale riguardo occorre ribadire alcuni punti fermi che vengono illustrati in un ordine del giorno che ho presentato affinché si impegni il Governo, nelle diversi sedi competenti e con atti coerenti con il diritto internazionale, a ribadire i princìpi relativi a materie concernenti la famiglia e la vita, che sono di competenza esclusiva degli Stati membri, le cui tradizioni costituzionali devono essere rispettate; a presentare in Parlamento la sua posizione prima dell'adozione di atti normativi comunitari che abbiano un impatto sul diritto e sulla famiglia; a proseguire, in coerenza con quanto avvenuto in sede di Convenzione europea, nell'impegno di introdurre le radici giudaico-cristiane nelle eventuali modifiche del Trattato di Costituzione europea, a partire dalla Dichiarazione di Berlino del prossimo 25 marzo. La revisione della Strategia di Lisbona ha ribadito il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese nella crescita e nell'occupazione, facilitandone l'accesso al VII programma comunitario. Merita di essere ricordato, inoltre, il problema dell'energia e la necessità di garantire sicurezza nell'approvvigionamento energetico ecosostenibile e competitivo, attraverso un piano di azione globale, in grado di assicurare migliore competitività del mercato interno dell'energia, la diversificazione delle fonti energetiche, la separazione effettiva delle attività di approvvigionamento dalle operazioni in rete. Non vanno sottovalutati i rischi per il mercato europeo della presenza di monopolisti mondiali. Tutto ciò, infatti, altera il funzionamento dei mercati, condizionati dalla crescente domanda mondiale, che crea instabilità sui mercati, e anche dai cambiamenti climatici.

costituisce un importante impegno della politica energetica europea, introducendo nuove strategie per rilanciare la competitività dell'Europa. Ma il nostro Paese, nel quadro della diversificazione delle fonti energetiche, non può né tralasciare né abbandonare l'opzione nucleare, tenendo conto dei più alti livelli di sicurezza ormai raggiunti. *(Applausi del senatore Possa).* Non dice nulla la spinta al nucleare di Paesi come l'Iran, grande produttore di petrolio, della Corea, dell'India e perfino, secondo notizie odierne, della Libia? Le recenti e gravi crisi di approvvigionamento hanno dimostrato la debolezza dell'Europa e i maggiori rischi per il nostro Paese; debolezza dopo la frammentazione dell'impero sovietico e proprio nel momento in cui questi nuovi Stati si sono misurati con le regole della concorrenza internazionale e con un sistema capitalistico ben lontano dalle regole del capitalismo democratico. Paradossalmente, il sistema politico sovietico garantiva maggiormente il rispetto dei contratti su una rete che si è poi frammentata. Sul problema dell'energia l'Europa non può muovere in ordine sparso, come si è purtroppo verificato, ma deve parlare con una sola voce, mettendosi in grado di competere unita rispetto alle nuove situazioni politiche, economiche e finanziarie. Si pongono anche obiettivi ambiziosi che riguardano le emissioni di gas serra, abbattendo le emissioni del 20 per cento entro il 2020, e le energie rinnovabili, che devono crescere dal 6 al 20 per cento per combattere i cambiamenti climatici. È stata data una risposta forte rispetto alle politiche energetiche e ambientali del futuro. Si apre una nuova fase, soprattutto per la ricerca, nella integrazione delle tecnologie, stimolando l'innovazione e la diffusione sul territorio, determinando benefici sulle attività produttive e sulle famiglie. Il clima non può essere considerato una componente invariabile per il complesso delle attività umane, ma diviene fattore variabile proprio in relazione alle azioni che l'uomo determina nella ricerca di sviluppo quale presupposto del successo sociale. Non è solo Kyoto il problema, ma anche una riconsiderazione delle infrastrutture inadeguate: mi riferisco sia alla tutela delle fasce costiere che alle opere di bonifica. Sarebbe necessaria una legge per un censimento della domanda pubblica in materia di sicurezza ambientale. Siamo all'avanguardia nelle applicazioni sulle osservazioni della Terra, sia con il progetto Galileo, sia con Cosmos-Skymed, che vanno finalizzati prevedendo protocolli sull'utilizzo dei dati. Il sistema del pianeta Terra è caratterizzato da un equilibrio che può subire alterazioni profonde a seguito di un aumento indiscriminato dei rifiuti inquinanti e da una modifica incontrollata degli elementi essenziali. Occorre allora rispettare i vincoli e limiti posti dalla natura per conservare l'equilibrio necessario. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, Bruxelles non deve essere vista solo come il luogo delle pagelle sui singoli Stati, come il luogo della produzione di sempre maggiore legislazione, di nuovi adempimenti burocratici, di nuovi oneri amministrativi, di nuovi sacrifici, ma come il luogo della semplificazione, della riduzione dei costi, dei maggiori vantaggi competitivi, delle nuove opportunità. È auspicabile maggiore partecipazione e consenso in luogo di un distacco crescente. Siamo impegnati nella ripresa del cammino europeo, riprendendo i riferimenti espliciti alle radici cristiane dell'Europa, un'Europa con una precisa identità culturale, un'Europa dei valori che non nasce da un relativismo senza princìpi, ma da valori che hanno plasmato l'identità europea nel corso dei secoli. Dobbiamo fare attenzione sui rischi di ulteriori allargamenti, se non vogliamo mettere a repentaglio la nostra identità. Guardare alle politiche per la famiglia con una nuova intensità significa ritrovare il coraggio di scelte forti, affermando i valori del patrimonio storico-culturale che è l'umanesimo cristiano europeo. L'Europa è chiamata a determinare un nuovo punto di equilibrio fra democrazia ed efficienza. Uscendo dalla crisi di crescita, l'Europa potrà diventare forte se sarà unita, se saprà parlare e dialogare con una voce sola, coniugando forza e ragione con nuove responsabilità, per tracciare nuove strade per nuove carovane, esportando cultura e idee. L'obiettivo della Carta costituzionale europea può significare una presa di coscienza e la ricerca della sua anima, di un'Europa come comunità di destino, come sostiene Edgar Morin, cioè di valori e non solo entità geografica. Certo, si può essere forti negli scambi commerciali, ma deboli nel disegno politico, nell'insufficienza delle istituzioni, nell'abdicazione continua alla storia e alle proprie radici. Noi guardiamo a costruire un'Europa politica da cui può venire la risposta ai problemi dei tempi nuovi, coniugando il culto dell'individuo e il culto della società, trovando nel nuovo umanesimo il giusto equilibrio tra progresso scientifico e progresso di valori morali e civili.

Signor Presidente, finalmente abbiamo la possibilità e l'opportunità di parlare di Europa in modo più disteso e compiuto. Questa è stata una scelta consapevole e un obiettivo perseguito dalla 14a Commissione credo che possa rappresentare anche una tappa verso un obiettivo che tutti condividiamo: far sì che le questioni dell'Europa si insedino permanentemente nella capacità di analisi e delle decisioni dei Parlamenti nazionali e quindi delle istanze rappresentative del nostro Paese. Il prossimo 25 marzo, Presidente, tra appena 12 giorni, saranno trascorsi 50 anni dalla firma del Trattato di Roma. Il dibattito che oggi si svolge in Senato a margine degli Atti comunitari nn. 7 e 8, relativi al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 e al programma di 18 mesi delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena, non può non risentire della vicinanza di quella data e del suo significato storico e simbolico; non può eludere un giudizio complessivo sul se e sul quanto l'Unione Europea sia riuscita a conquistare, in questo mezzo secolo, l'interesse dei suoi cittadini, divenendo nella concretezza e nella percezione comune uno strumento di miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei suoi abitanti; una domanda a cui nessuno può sfuggire, signor Presidente e signor Ministro. Nonostante i traguardi raggiunti ed il suo consistente allargamento territoriale, permane ancora (credo occorra dirlo senza giri di parole o sottintesi) un divario tra le domande che emergono dal profondo del corpo sociale, dalla materialità delle condizioni dei popoli che la compongono e l'impegno complessivamente ultraliberista della costruenda Unione Europea, che assume come direttrice portante la competitività e su questo altare spinge verso la consegna al mercato di servizi pubblici, anche di quelli ad alto contenuto sociale, ripete il *refrain* sulla riforma delle pensioni, una riforma naturalmente peggiorativa, che rischia di aggravare le condizioni già pesanti per molti lavoratori che hanno superato l'età del lavoro. L'*impasse* che si è prodotta nel percorso di ratifica del Trattato costituzionale ne è, dal nostro punto di vista, la prova più evidente ed evidente è la reale natura della crisi segnata dalle bocciature referendarie di Francia e Olanda e dal silenzio-dissenso di molti altri Paesi. Un dato che non possiamo eludere e che va letto per quello che è: il risultato di una sostanziale ambiguità tra un processo costituzionale che, per essere tale, avrebbe dovuto muovere dal riconoscimento di una comunità di destino - come qualcuno ha detto - e dalla conseguente partecipazione democratica basata sul suffragio universale e la natura invece di un Trattato, come tale siglato dagli Esecutivi dei Paesi membri sui contenuti materiali delle politiche europee. Un'ambiguità, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, racchiusa nello stesso artifizio della sua definizione di Trattato costituzionale, dove troppo deboli sono i diritti, in molti casi arretrati rispetto al diritto nazionale dei Paesi membri, e troppi forti le scelte politiche contenute nella terza parte, tali da renderle quasi indisponibili alla sovranità del Parlamento. Nello stesso programma globale di cui oggi discutiamo, la Presidenza tedesca si impegna a presentare una relazione al Consiglio fondata su ampie consultazioni con gli Stati membri, passando poi il testimone alle altre due Presidenze purché «le iniziative necessarie siano prese nella seconda metà del 2008 al più tardi» quasi ad evitare ogni possibile intreccio tra un percorso a basso tasso di democrazia indiretta, come quello fino a qui proposto, con l'appuntamento invece ad alto tasso di democrazia diretta costituito dalle elezioni europee del 2009. Noi crediamo, invece, che da quell'intreccio potrebbe determinarsi l'uscita dall'*impasse* che riconsegni l'Europa ed il suo futuro ai suoi cittadini, riattivando partecipazione e consapevolezza. Una critica, come vedete, dura e radicale, ma che non ci induce verso approdi euroscettici, verso particolarismi nazionalistici, e anzi ci fa continuare ad essere caparbiamente euroconvinti, ad individuare con forza la sfida europea come il gorgo entro cui si può e si deve lavorare per un altro mondo possibile, a cominciare da un'altra Europa possibile. Nessun fenomeno politico e istituzionale è monolitico, impermeabile alle richieste ed alle spinte che provengono dalla società reale. Nessuna autonomizzazione della realtà può proporsi come assoluta e definitiva. Dentro quel gorgo siamo a cogliere ogni elemento di positiva novità, a raccoglierlo ed a spingerlo verso un possibile ulteriore avanzamento. Nuove richieste e nuove esigenze, pure in un quadro dove permangono contraddizioni ed a volte arretramenti, nuovi paradigmi, nuove parole, nuove istanze avanzano sullo scenario di quella che qualcuno ha voluto definire con disprezzo la vecchia Europa. Con questo spirito abbiamo apprezzato come un elemento di forte e positiva novità la missione in Libano, a cui il nostro Paese ha dato un contributo decisivo, e l'impegno in quell'area verso un'ulteriore possibile stabilizzazione, necessaria a contrapporre al conflitto mediorientale una soluzione di pace basata sul traguardo del riconoscimento di due popoli e due Stati. Vi è, signor Presidente, un positivo richiamo all'esigenza di sviluppare la cooperazione internazionale, in particolare l'inserimento nelle priorità, così come recita il programma, del secondo vertice UE-Africa che dovrà svolgersi sotto la Presidenza portoghese, e un vertice UE-America Latina sotto la Presidenza slovena. In questo quadro di apertura il nostro Paese può avere un ruolo centrale nelle relazioni con l'area del Maghreb, recuperando la tradizionale direttrice di politica estera messa in secondo ordine nella passata legislatura. Abbiamo anche apprezzato gli obiettivi declinati dalla Strategia di Lisbona: la creazione di lavoro buono, lo sforzo di coesione sociale, la valorizzazione delle risorse umane, dell'ingegno e dei saperi, se pure segnati ancora dal permanere di equivoci di fondo, da una subordinazione di tali obbiettivi alle logiche finanziarie, all'idea del mercato come solo elemento sovraordinatore capace di determinare ed orientare i processi sociali, da un'idea del lavoro come esclusivo strumento di produzione, non come fattore fondamentale del diritto, come fattore identitario di inclusione sociale e segnato così dalla flessibilità come elemento ineludibile, come destino ineludibile, velato dall'utilizzo dell'ossimoro della «flessicurezza». Così la costruzione di una nuova politica energetica, elemento centrale, io credo, da valutare positivamente nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, richiamata nel programma dei 18 mesi, sviluppata nelle comunicazioni nn. 11, 12 e 13 della Commissione e sostanzialmente confermata nella riunione dell'ultimo Consiglio europeo. Ma anche qui, mentre finalmente si affronta la questione della sostenibilità ambientale e del riscaldamento del pianeta, c'è bisogno di pesare i costi dell'azione e dell'inazione, pure in una serrata analisi disvelante (come quella del rapporto Stern), come se il dovere della solidarietà verso la generazioni future, a cui non possiamo lasciare in eredità un disastro ambientale, fosse limitato al risultato di un'operazione matematica in cui si sommano e si sottraggono punti di PIL. Certamente la questione energetica è essenziale per rilanciare il ruolo dell'Europa sul teatro internazionale, ma la ricerca di nuove tecnologie nella produzione di energia da fonti rinnovabili a bassa o nulla emissione di carbonio non è solamente un'opportunità economica, una nuova merce a forte valore aggiunto che può rispondere alla domanda di Paesi in tumultuosa crescita economica che può trovare lì un collocamento economico. Dentro questa parzialità ed insufficienza del punto di vista sta il tentativo di percorrere strade che che solo in apparenza sono nuove, come la promozione di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica, che ripropongono invece problemi già conosciuti sull'accumulo di scorie di cui non si è ancora in grado di prevedere impatto e gestibilità ambientale. Non è solamente attraverso gli scambi attivi e i guadagni d'impresa che questo nostro continente può rilanciare il proprio ruolo ma anche, e io credo soprattutto, attraverso la costruzione di modelli socialmente ed ambientalmente compatibili, che non stiano in piedi solamente in virtù di un successo competitivo ma che siano in grado di proporre un modello generale di nuovo umanesimo. Verso questo obiettivo può avanzare un'Europa dei popoli, della pace, del lavoro, dei diritti, della differenza di genere, capace di parlare alle menti ed anche al cuore dei suoi cittadini, non chiusa in se stessa, ma aperta alla costruzione di un nuovo mondo possibile e sempre più necessario. È questo, per noi, il modo migliore di interpretare la celebrazione della ricorrenza del prossimo 25 marzo, nelle sue iniziative istituzionali ai più alti livelli e nelle sue articolazioni territoriali.

«L'Europa non esiste; bisogna crearla». È passato molto tempo da quando uno dei padri dell'Europa, Jean Monnet, pronunciava queste parole, e l'Unione Europea è una realtà. Risultato di un lungo processo di integrazione culturale e sociale, figlia della civiltà classica e della tradizione giudaico-cristiana, del Rinascimento e del Secolo dei Lumi, l'Europa che si è andata delineando negli ultimi anni è molto diversa da quella emersa agli esordi o ancora nei decenni scorsi. Il cosiddetto *big* *bang*, l'allargamento ai nuovi Stati membri, ha infatti portato con sé un radicale mutamento degli scenari. Si potrebbe quasi dire che l'Europa del futuro è più vicina a quella del secolo scorso, costituita da una pluralità di razze, lingue e Paesi, che a quella immaginata dai suoi padri fondatori. Il lungo processo di integrazione economica e l'introduzione dell'euro hanno avuto certamente un ruolo aggregante in termini monetari, mentre l'integrazione politica è ancora di là da venire. La sfida cui siamo chiamati oggi è quella di dare vita a un'Europa vicina ai cittadini, a un'Europa dei popoli oltre che a quella degli Stati. Se è certo, infatti, che l'Unione è riuscita a divenire un'istituzione unica nella storia dell'umanità, non sempre essa è riuscita a toccare il cuore e lo spirito di coloro che ne fanno parte. La domanda che tutti dovremmo porci è: cosa vuole dire oggi essere europei? In un complesso mosaico di Nazioni e popoli, quale è l'Europa, diventa sempre più difficile cogliere un'identità comune e un *idem* *sentire* se non si collega a radici lontane, unificate e attualizzate da una comune prospettiva del futuro. Ciascuno deve dare il suo contributo ad edificare l'Europa che verrà, costituita da molti Paesi, tra loro diversissimi, in cui i rischi di dispersione e scarsa partecipazione si fanno sempre maggiori. Se è vero, come diceva il presidente Jacques Delors e come ha ribadito Angela Merkel, che l'Europa «deve avere un'anima o, meglio, trovare la sua anima», bisogna altresì tenere conto del fatto che quella Europa potrebbe avere ben più di un'anima e che il futuro è rappresentato dalla capacità di incanalare le diverse anime in un unico flusso, selezionando quanto c'è di meglio in ognuna di esse. Occorre ribadire ancora una volta, onorevoli colleghi, che l'Europa è nata su un disegno economico e non politico; la cooperazione monetaria avrebbe dovuto rappresentare solo un aspetto, anche se centrale, di un processo molto più ampio di integrazione produttiva e disegno di un sistema capace di imporsi in una logica transnazionale. Così non è stato. Dopo la fase agricola degli anni Cinquanta e Sessanta e quella industriale dei decenni passati, la sfida è ora nella costruzione dell'Unione neoindustriale del nuovo millennio. Sono alle nostre spalle le due Europe che avevano unificato il progetto economico-comunitario. Dopo l'Unione del carbone e l'acciaio, dopo la battaglia per le quote latte e per il burro, è venuto oggi il tempo dell'Europa delle reti; bisogna ritrovare, signor Ministro, forti motivazioni ideali che fungano da fattore aggregante per la costruzione europea o rischieremo solo di mantenere in vita un'Europa degli interessi che non sa parlare a quella dei cittadini, che non sa coinvolgere emotivamente le coscienze, che è solo in grado di evocare sacrifici economici non controbilanciati da contropartite emotive. Integrare le diversità culturali, economiche e sociali dell'Europa per costruire la nuova civiltà dei valori è un compito irrinunciabile della nostra politica. Fatta l'Europa - per parafrasare un'altra frase celebre - occorre fare gli europei. In questo quadro e con queste doverose premesse, ho trovato corretta la risoluzione approvata dalla Commissione politiche dell'Unione Europea, pur dovendo constatare che, per l'ampiezza dei temi trattati e la complessità di ciascuno di essi, sarà opportuno concentrarsi su elementi concreti che realizzino effettivamente quanto ci si propone.

Democrazia, libertà, progresso economico, coesione e solidarietà sociale, rispetto ambientale: tutti temi importanti, complessi, che sono alla base della nostra idea di Europa, ma che poi - chissà perché - stentano a tradursi in un linguaggio comprensibile ai cittadini, che tocchi il loro cuore e la loro anima, oltre che il loro portamonete. Guardo con profondo interesse al programma legislativo e al lavoro della Commissione europea per il 2007, che cerca di far fronte alle attese dei cittadini e alle sfide della globalizzazione, del cambiamento climatico, del problema energetico e del terrorismo. Reputo assolutamente positivo il fatto che siano state definite delle azioni concrete, le 21 iniziative strategiche per dare un reale seguito a tante buone intuizioni, accompagnate da 60 iniziative prioritarie. Ribadisco però che, in mezzo a tanti temi elevati e di gran valore, due concetti bisogna tenere bene in mente; concetti che devono animare ed indirizzare le nostre azioni. Da una parte, a livello più teorico e ideale, c'è la sfida per l'identità: solo comprendendo chi siamo possiamo avere elementi certi su dove andare. Troppo spesso dell'Europa si continua ad avere una visione per metà fideistica e per metà retorica. Quello che all'inizio è stato elemento di forza e di costruzione dell'Unione, cioè la sua focalizzazione sull'economia, diventa oggi una debolezza; mentre in altri campi essa rischia di esprimere miti e valori inadeguati al suo ruolo internazionale e alla sua struttura. Il rischio, infatti, è che la tolleranza dell'Europa diventi solo retorica, le politiche sociali siano poco consistenti, la disponibilità ad affrontare sacrifici necessari per la gestione, lo sviluppo e l'affermazione internazionale di un immenso numero di persone sia inesistente. Non vorrei che, oltre agli aspetti economici e di mercato, l'unico denominatore comune dell'Europa siano gli egoismi individuali, regionali e nazionali. Occorre dunque dar vita ad un vero patto per l'Europa (questa è la nostra proposta), in cui Stati nazionali, burocrazie, imprese ed associazioni siano parte integrante e trainante: questa è l'Europa che immaginiamo. Da una parte, a livello più pratico, occorre attuare con forza in Italia la Strategia di Lisbona, poiché siamo decisamente in ritardo rispetto agli obiettivi da raggiungere nel 2010. Alcuni dati, forniti da «Il Sole 24 ORE», potranno essere esemplificativi di quanto dico. Il tasso di occupazione in Italia dovrebbe essere al 70 per cento, ed è al 58; certamente molto è stato fatto, con la legge Biagi del precedente Governo, ma c'è ancora una lunga strada da percorrere. La spesa in ricerca e sviluppo è all'1 per cento; dovrebbe essere al 3

Tutto questo, signor Presidente, fa capire quanto importante sia, all'interno del dibattito che la Commissione ha svolto sulla base dei due documenti programmatici europei, sul tema delle riforme istituzionali e sulla campagna di sensibilizzazione su ragioni e valori dell'integrazione europea nel Paese, dare il giusto rilievo e le corrette spiegazioni anche all'attuazione della Strategia di Lisbona. Pur ribadendo il mio accordo alle iniziative strategiche e prioritarie che la Commissione vuole adottare (dalla modernizzazione dell'economia al riesame del mercato interno, dall'eliminazione delle barriere nel mercato del lavoro al puntare sulla «flessicurezza», dalla migliore gestione dei flussi migratori all'analisi strategica in materia di energia, dal miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei al rinnovo della strategia per accesso al mercato e così via), non posso che dichiararmi perplesso per l'assoluta assenza, anche nella nostra risoluzione, signor Presidente, di un qualunque accenno a politiche euromediterranee.

l'Europa aveva compreso quanto fosse importante impegnarsi attivamente per lo sviluppo del Mediterraneo poiché esso è garanzia indispensabile per garantire pace, sicurezza e prosperità in tutta l'Unione. La Prima Conferenza euromediterranea tenutasi a Barcellona nel 1995 aveva deciso in modo impegnato una strategia ambiziosa e a lungo termine di partenariato euromediterraneo, delineata nel Documento conclusivo della Conferenza, la Dichiarazione di Barcellona, e nell'allegato Progetto di lavoro. Gli obiettivi principali della nostra politica euromediterranea erano: la creazione di una zona di pace e stabilità politica; la nascita di un'area di prosperità economica comune da realizzarsi mediante l'implementazione della politica del libero scambio fra i Paesi del Mediterraneo, fino alla creazione di una più vasta zona di libero scambio entro il 2010; l'implementazione del dialogo, della comprensione e della tolleranza fra i popoli della Regione. Un approccio globale, insomma, con un partenariato diviso in tre settori definiti i «tre pilastri del processo di Barcellona».

Occorre creare una rete di infrastrutture materiali fra loro collegate che consentano circolazione di merci e di persone, e infrastrutture immateriali quali codici, scuole e istituzioni. Bisogna, soprattutto, compensare lo scivolamento dell'Europa verso Est realizzato grazie a calcoli economici che mettono la Germania al centro, e da cui noi rischiamo di essere tagliati fuori. Troppo spesso siamo - o vogliamo essere - alla periferia dell'Impero. Guardo con preoccupazione a questa Europa che si disegna sempre più attorno all'Atlantico e sempre meno al Mediterraneo. Il posizionamento geografico del nostro Paese la sua storia, signor Ministro, ne fanno un ponte fra Nord e Sud del Mediterraneo e una formidabile opportunità strategica, se colta in tutte le sue implicazioni e gestita in chiave di politica industriale. È l'Italia, dunque, che ha il dovere di investire nel patrimonio mediterraneo pensando ad un Patto europeo che incentivi modelli di sviluppo ecosostenibili, dando vita a progetti infrastrutturali, energetici, turistici, ambientali capaci di delineare a Sud un sistema integrato per 500 milioni di persone. Credo che questo debba essere un elemento fondamentale nella nostra politica, ora e in futuro. Mi auguro che il prossimo appuntamento delle celebrazioni del 50° anniversario dei Trattati di Roma - che si terrà non a Roma, ma a Berlino, per l'appunto possa servire a ribadire non solo la molta strada percorsa, ma anche quella che resta da fare e, soprattutto, la direzione in cui farla. Se non riusciremo nei nostri obiettivi, andremo incontro a rischi sia nella costruzione europea che nel sistema Italia: nella costruzione europea perché oltre l'enfasi e la retorica ci sarà il vuoto e si renderà l'Europa più lontana e non più vicina al cuore dei suoi componenti e ancora meno comprensibile; nel sistema Italia - e concludo perché questo, fatalmente emarginato da un asse Est-Ovest e non più Nord-Sud, non sarà in grado di cogliere le grandi opportunità oltre che i costi che da quella Europa derivano. Partecipare in modo paritetico, in diritti e doveri, all'Europa del futuro è la missione a cui è di fronte l'Italia, l'unica possibile per il suo sviluppo.

credo ci troviamo di fronte ad un'opportunità davvero formidabile, cioè quella di parlare di Europa in modo così compiuto e totale nel momento in cui ci accingiamo a celebrare i primi 50 anni di vita, di attività e di attualità dei Trattati di Roma. Sappiamo benissimo che la grande intuizione di un accordo a livello europeo avvenne nel 1951 quando nacquero la CECA e l'EURATOM, le prime forme di cooperazione a livello europeo. Ora quei giorni, quelle date e quegli eventi, messi a confronto con lo spirito con il quale ci accingiamo a celebrare gli avvenimenti stessi, a volte sembrano quasi stridere; si ha quasi l'impressione che vi fosse più entusiasmo e più concretezza allora che non in certi interventi oggi svolti sui temi europei. temi europei. Credo che una vera celebrazione debba guardare sempre e comunque avanti. La storia ha fatto il suo percorso e oggi il traguardo avanzato, dopo avere raggiunto negli ultimi dieci anni tre formidabili grandi riforme storiche, è quello della Costituzione europea. Negli ultimi dieci anni, chi ha vissuto l'esperienza in Europa ha avuto l'opportunità di celebrare la nascita dell'euro, che - lo ricordiamo - non fu una realizzazione del 2002 quando ottenemmo concretamente in tasca le monete, ma fu una sofferta scelta del 2 maggio 1998 quando nacque la moneta virtuale.

per cui anche la Costituzione non debba diventare la nostra misura comune con cui confrontarci nel futuro. Il modo migliore per celebrare il dei Trattati di Roma sarebbe quello di dare uno slancio, un rilancio convinto ed importante, proprio al Trattato costituzionale. Al riguardo, vorrei soffermarmi perché indubbiamente è il traguardo al quale dobbiamo puntare senza troppe teorie,

Innanzi tutto il Consiglio europeo, composto da Capi di Stato e di Governo, diventerà un'istituzione stabile, con un Presidente in grado di rappresentare l'Unione nel suo complesso e per un periodo più lungo di quei sei mesi che stavano trasformando

invece un'istituzione dotata di una Presidenza stabile, che potrà giocare un ruolo più incisivo di impulso, di indirizzo e di guida politica dell'Unione confacente alla sua composizione ed al suo rango. Si tratta di un ruolo che il Consiglio europeo ha svolto finora

il Consiglio dei ministri dell'Unione, un'istituzione che rappresenta gli Stati membri, avrà una struttura organizzativa nuova, dove saranno chiarite e distinte le funzioni legislative da quelle di azione politica, in particolare per quanto concerne la politica estera, la politica economica e la politica della giustizia, cioè la possibilità di avere una Presidenza stabile che darà anche al Consiglio una maggiore continuità d'azione, soprattutto in materia legislativa. Grande interesse e grande attualità in questi giorni ha quanto l'Europa si accinge a inventare, diciamo così, ma sulla base concreta della Costituzione,

che riuscirà, se realizzato, se dotato anche della fiducia e degli strumenti necessari, a rappresentare l'Europa in maniera autorevole, finalmente, sullo scenario internazionale.

approvato del Parlamento europeo, non succederà nulla. Il Parlamento europeo, che invece rappresenta direttamente l'Unione, con la Costituzione diventa legislatore a pieno titolo, accanto al Consiglio dei ministri, ed è chiamato tra l'altro a nominare la Commissione europea. la Commissione vedrà anche rinnovato il suo ruolo in un equilibrio istituzionale tutto nuovo e tutto da applicare, ed è una novità importante: essa diventa un'istituzione politica, non più soltanto amministrativa o paragovernativa. Il suo Presidente non sarà più un *primus* *inter pares* ma un vero e proprio Presidente, dotato di poteri di indirizzo e di coordinamento; sarà designato sì dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata ma poi deve essere accettato dal Parlamento europeo, che terrà conto anche della proporzionalità politica che si è verificata nelle ultime elezioni europee. Con la Costituzione la Costituzione europea non cambieranno soltanto le istituzioni ma cambieranno soprattutto le politiche. La politica estera e di sicurezza comune, cui ho accennato prima parlando del nuovo attore che la rappresenterà in Europa, nel progetto di Costituzione, unifica, sotto uno stesso titolo, l'insieme delle relazioni esterne, dotando di coerenza e continuità l'azione stessa e rafforzando gli strumenti della protezione esterna dell'Unione. In materia di politica estera e sicurezza comune, il fatto più rilevante è proprio la creazione di un Ministro che si chiamerà finalmente così; mediante la formula del doppio cappello, il Ministro degli esteri rappresenterà il Consiglio e anche la Commissione, in quanto diventerà automaticamente Vice presidente della Commissione europea. alla politica di sicurezza e di difesa, tutti sappiamo quanto vi sia bisogno di questo coordinamento; una politica comune di difesa è necessaria se vogliamo sviluppare una politica estera di sicurezza comune dotata di un minimo di credibilità. La proposta prevede le cosiddette cooperazioni strutturate e la cooperazione più stretta; ancora una volta, si dà la possibilità ai Paesi membri di non stravolgere i propri orientamenti di base. Le prime consistono in gruppi di Stati membri con la volontà di assumere impegni vincolanti in materia di capacità militari; la seconda è una clausola di mutua difesa, sullo stile dell'articolo 5 del Trattato di Bruxelles, che costituisce l'Unione Europea di difesa. grande attualità è anche lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che raccoglie tutte le istanze dei cittadini europei, per esempio in materia di cittadinanza e di immigrazione. e di immigrazione. Questo spazio viene consolidato con l'estensione del voto a maggioranza qualificata e della procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo. Il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e penale costituisce la base di un vero spazio giudiziario europeo. Il progetto di Trattato, infatti, incorpora l'embrione di un ordine pubblico europeo. Abbiamo discusso e parlato a lungo di istituzioni e istituti come Eurojust ed Europol, forse mai compiutamente realizzati, anche perché ogni volta incontravano, come l'istituto della procura europea, le remore, le prudenze e diciamo pure l'opposizione di certi Paesi membri non disposti a concedere nulla della propria sovranità su tale territorio. Il Trattato, grazie anche al Trattato di Nizza e alla Costituzione, offre grandi e nuove garanzie per i cittadini sotto ogni forma di vita. Si è realizzata la famosa Europa dei cittadini che si vaticinava al tempo del Trattato di Maastricht e che oggi è una realtà proprio grazie a Nizza. Nel quadro della lotta contro il crimine organizzato, il terrorismo e il traffico di esseri umani, la Costituzione concede e attribuisce alla politica di libertà, sicurezza e giustizia grandi opportunità. Ad esempio, in tale settore è prevista la misura del congelamento di fondi e di titoli appartenenti a persone fisiche o giuridiche macchiatesi di delitti in questo campo. La disposizione colma una lacuna che esisteva nei Trattati attuali, che prevedevano che si potessero congelare i beni di terroristi, di sfruttatori della prostituzione e di trafficanti di esseri

il tema della *governance* economica vede la Commissione incrementare notevolmente le proprie competenze e le proprie possibilità con il coordinamento delle politiche economiche e il controllo dell'adempimento di procedimenti come, ad esempio, quello dell'eccessivo L'adozione sul piano esterno di misure a maggioranza qualificata o su proposta della Commissione consente alla stessa Commissione europea di avere un ruolo di maggiore orientamento della politica economia e monetaria dell'Unione Europea. Il grande tema, che è ancora latitante anche nella Costituzione, è quello della politica fiscale. Anche qui, grandi e lunghi dibattiti, ma in tema di politica fiscale l'egoismo - lasciatemelo dire - di taluni Paesi membri non ha consentito alcuna forma di armonizzazione, parola che suonava addirittura ostile e ostica per tutti coloro che difendevano, viceversa, le politiche fiscali nazionali. Continuerà quindi ad un settore, una branca dell'economia, decisa all'unanimità in seno al Consiglio, con la consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Il Trattato prevede comunque, per alcune disposizioni, forme di cooperazione in tema fiscale: questo è il massimo, a quanto pare, della comunione di idee e di intenti oggi possibile. Per concludere, anche oggi stiamo parlando della Costituzione con qualche dubbio, qualche remora e motivo di dibattito. Probabilmente se ne parlerebbe ancora hanno fatto i cosiddetti padri convenzionali a un certo punto a tagliare corto. Dopo diciotto mesi di confronto, chissà con quali sofferenze (le possiamo immaginare perché li vedevamo quotidianamente alle prese con questo difficile compito) e mille votazioni, mille confronti e dibattiti, vedo qui un emendamento che ripropone ancora l'antico tema delle radici cristiane per il quale almeno la mia parte si è battuta fino a diventare pateticamente martire in un ambiente ostili. A tal proposito, si è girata la polpetta in ogni direzione: le radici cristiane, poi le cattoliche, le cristiano‑giudaiche, ma non si è arrivati a nulla. A questo punto, un emendamento certamente lo voteremo, ma avrà il significato simbolico di una pia utopia sacrificata chiaramente e inevitabilmente sul piano del pragmatismo degli altri Stati. Non dimentichiamo che il il processo di integrazione europea ha delle regole e si muove secondo logiche diverse dai processi di integrazione dei diversi Paesi. Non a caso, uno dei grandi padri dell'Unione Europea, Jacques Delors,

l'unione economica dell'Europa, il vero mercato unico, le vere regole condivise per quanto riguarda la convivenza sui mercati, Jacques Delors non è riuscito a dare altrettanta concretezza ed incisività alle politiche rivolte ai cittadini,

riscosso da nessuno. L'Europa non avrà mai un unico popolo, non esisterà mai un popolo europeo bensì popoli diversi uniti da un comune destino.

In un'Europa sempre più diversa, con popoli sempre più diversi che ancor più difficilmente, rispetto a quando eravamo 12 o 15 membri, troveranno motivi di coesione, è ancora più attuale il

una previsione con una frase che mi piace ripetere.Egli affermò: «La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche». sostenendo: «L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto».

la sua struttura di previsione mai compiuta, ancora attuale e sulla quale c'è ancora molto da lavorare. Spero davvero che il 25 marzo, in occasione delle celebrazioni, si sappia cogliere il significato di questa frase senza fermarsi ad una celebrazione storica e retorica o alla ripetizione di concetti già manifestati, ma si sappia evidenziare ed interpretare la forza e il significato, soprattutto profetico, di un'idea che ancora oggi, nonostante gli sforzi, non si è realizzata compiutamente.

delle ultime decisioni assunte dall'Unione Europea. Da un lato, vi è il programma della Commissione che si connota di 21 iniziative strategiche ben precise; poi il fatto che non vi è più il Piano strategico triennale del Consiglio, che si sostanziava del Piano operativo annuale, ma un programma concreto di 18 mesi, che mette insieme le tre Presidenze. In questo modo infatti il raccordo è più agevole e ne scaturisce una più facile individuazione di obiettivi concreti. Non è certo possibile affrontare compiutamente i diversi punti sottoposti alla nostra attenzione, ma volendo racchiuderli in uno sguardo di sintesi partirei da quella che mi sembra la vera novità prodottasi negli ultimi interventi dell'Unione Europea, quella che ritrovo nel discorso che Angela Merkel ha tenuto, introducendo la presentazione del programma dei 18 mesi; una novità che non attiene ai meccanismi di Governo, bensì ai fondamenti ideali che ne guidano l'azione. Mi riferisco in modo specifico al richiamo che la Merkel ha fatto ad un'affermazione di Delors, nella quale dice esplicitamente: «l'Europa deve tornare a darsi un'anima»; poi si corregge e dice: «deve trovare la sua anima». Sembra un pensiero poco concreto e un po' romantico. In realtà la Merkel ha posto l'accento sul vero problema: la crisi che avvolge l'Unione Europea è tutta infatti riconducibile all'appannamento dei moventi, delle ragioni ideali del suo percorso, in mancanza delle quali ogni azione delle istituzioni comunitarie si connota ineluttabilmente di quel grigiore burocratico che tiene lontani i cittadini europei da quel mondo, quel mondo, che pure costituisce la fonte più copiosa del proprio futuro. La Merkel questo lo intuisce, ma dà una risposta non all'altezza della sua stessa domanda: la tolleranza infatti non può essere l'anima dell'Europa; essa è una delle sue caratteristiche, un modo di guardare la storia dell'umanità, i rapporti con gli altri. L'anima da trovare sta nel recuperare la missione dell'Europa, alla luce sia dei valori in nome dei quali si è sviluppata l'integrazione, sia dei nuovi segni dei tempi, che gradualmente consentono a chi sa e vuole leggerli di rimodulare il proprio percorso con sempre maggiore consapevolezza dei traguardi. Ho apprezzato gli interventi sia di Santini sia di Baccini. Ma attenzione: non possiamo affermare, caro collega Baccini, che i nostri padri hanno pensato all'inizio ad una Comunità Europea che avesse una natura soltanto economica. Nei discorsi di De Gasperi, già nel 1946, è chiara la necessità di un esercito europeo, che è futuro rispetto a noi, e vi era la piena consapevolezza della dimensione politica dell'Europa, anche se i primi passi dovevano inevitabilmente e necessariamente avvenire attraverso l'integrazione di tipo economico. Ma è proprio questo il segno della crisi che noi attraversiamo: il vertice straordinario, convocato per celebrare il cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma, non dovrà - spero - solo ribadire genericamente la vocazione politica e non soltanto economica dell'Europa, ma tracciare nuovi orizzonti al suo cammino. cammino. Quando i nostri Padri iniziarono il processo di integrazione, avevano immediatamente alle spalle una pagina apocalittica della storia dell'umanità, forse la più tragica, quindi l'unità dell'Europa fu sentita soprattutto come una scelta che scongiurasse definitivamente il ripetersi di simili scenari. Ma oggi l'unità dell'Europa deve trovare una sua nuova ragione e una sua nuova anima nel rapporto con il pianeta, con il mondo. La globalizzazione tutti la definiscono come sfida, come fosse un nuovo Golia da vincere; invece essa è, a mio avviso, un passaggio di grande crescita dell'umanità, perché ci consente di vivere i processi umani e politici come cittadini del mondo. Essa si pone come una risorsa di coscienza collettiva, di nuova e moderna consapevolezza che tutta l'umanità è, in fondo, una comunità di destino. Come si può non vedere che è proprio in queste coordinate che l'Europa deve trovare la sua anima? Abbiamo sempre pensato che l'Unione Europea servisse solo agli europei e avesse un senso solo per loro. Oggi invece siamo nelle condizioni di comprendere che l'antica Europa, se unita e aperta, è una giovane promessa per il mondo intero, perché è nelle condizioni di innervare gradualmente nella convivenza umana, senza tentazioni egemoniche, politiche o culturali, quei princìpi di solidarietà, libertà, tolleranza, rispetto delle diversità e pace di cui il mondo ha assolutamente bisogno. Questa mi appare oggi la missione dell'Europa, questa la sua anima. Se proveremo a collocare dentro questo orizzonte tutte le questioni aperte e irrisolte che l'Unione porta con sé, dal nuovo Trattato costituzionale all'ambiente, dall'energia ai limiti dell'allargamento, presto ci renderemo conto che avremo delle risposte facili, come sempre avviene lungo un percorso se la meta è chiara e agognata. Come non ritenere segni dei tempi l'impotenza delle istituzioni territoriali e nazionali dinanzi a questioni come quelle dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza? Come non vedere che se la politica non allargherà i suoi orizzonti dotandosi di istituzioni sempre più rappresentative su alcuni temi, fino ad arrivare a essere planetarie, temi, fino ad arrivare a essere planetarie, essa decreterà la sua definitiva inutilità, sancendo con la propria morte quella della democrazia? In queste prospettive dobbiamo anche ripensare a come rendere quanto prima operativo il Trattato costituzionale; senza un'Unione più integrata, unita e capace di decidere sarà infatti impossibile aprire quella che io chiamo la seconda fase dell'integrazione europea, quella che guarda ai rapporti con il mondo. Ciò che è mancato intorno al Trattato costituzionale è stata proprio la tensione ideale verso questi nuovi traguardi. Credete che i francesi e gli olandesi, fondatori della Comunità Europea, siano diventati all'improvviso antieuropeisti? No, i risultati di quei *referenda* sono stati il segno e il frutto di un'elaborazione del Trattato costituzionale tutta chiusa nei tecnicismi normativi, priva di una tensione politica e di un pensiero lungo sul destino dell'Europa. Non possiamo non ricavarne una lezione importante. Riprendiamo dunque con forza le ragioni profonde del progetto Europa.

il testo della risoluzione, però mi sembra così povero. Scusate la franchezza, ve lo dico con molta umiltà, senza alcuna supponenza, per carità. Il 25 marzo abbiamo un'occasione solenne per tentare di mettere sotto gli occhi dell'opinione pubblica europea il bisogno disperato di profezia che ci Con le regole, i buoni propositi, le buone pratiche e senza un grande slancio, una grande tensione ideale il processo di integrazione, la missione, quell'anima di cui parlava la Merkel, non la ritroveremo più.... *(Brusìo).* Vi chiedo scusa, per cortesia, è un argomento che dovremmo cercare di sentire un po' di più, perché se questo deve essere il livello dell'attenzione che il Parlamento rivolge a questo tema è estremamente sconfortante. sconfortante. Abbiamo la fortuna di avere oggi qui il Ministro. Signor Ministro, dobbiamo crederci, e lei ci crede più di me, ma in questa occasione, che si presenta semplicemente come un'occasione celebrativa,

concluse un suo memorabile intervento al Parlamento europeo con queste parole: «Non dimentichiamo mai che l'unione dell'Europa è azione dello spirito». Questa è la nostra unica forza. Ognuno di noi può avere proprie idee su come la storia procede: chi guarda alla Provvidenza, chi alla casualità, chi crede che vi sia un'anima della storia, ma non possiamo negare che davanti ai grandi segni dei tempi siamo chiamati ad un supplemento d'anima, in mancanza del quale nulla ci ridarà l'attenzione verso l'Europa che oggi non è più una questione che riguarda gli europei, ma il mondo intero. È questa nuova consapevolezza che ci può dare la forza di una nuova missione e di una nuova anima. Dunque, concludo dicendo che solo questo slancio ci potrà far superare le attuali difficoltà e ci potrà consentire di riprendere a camminare insieme come europei, incontro al mondo intero. Può sembrare una nuova utopia, io lo confermo in pieno: è così. Tommaso Moro, un padre della nostra Europa, ci ricordava qualche secolo fa che senza utopia si vive, ma non si costruisce la storia.

ma è abbastanza contraria al tipo di Europa che è stato forgiato in questi anni dalle istituzioni comunitarie. La Lega Nord da sempre si batte per un'Europa dei popoli, rispettosa delle diversità e realmente democratica; per questo rifiutiamo l'approccio superficialmente ottimistico e il fideismo acritico che permeano i discorsi politici quando si parla di Europa. Oggi, l'Europa è una costruzione senza identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini; un'istituzione in cui il potere è accentrato e gestito in modo elitario, un modello che esaspera gli aspetti negativi dello Stato centralizzato (una sorta di super Stato) senza dare risposte tangibili alle richieste che vengono dalle periferie. un esempio su tutti, basterebbe chiedere ai 400 o 500 milioni di cittadini europei se sanno cosa è la Commissione.

In realtà, l'Europa in questi anni è stata gestita dalla Commissione europea, che è tutt'altra cosa, e non è eletta dal popolo, ma è nominata dai Governi delle varie

concetto e che ancor meno lo abbiano compreso fino in fondo. Un'Europa così strutturata non può essere forte e coesa per affrontare da protagonista l'arena internazionale; continuerà ad aumentare la sua fragilità e la sua conflittualità interna se si proseguirà senza un profondo rinnovamento e un cambio di rotta e se si continuerà ad insistere nell'allargamento ad altri Stati, come la Turchia, troppo lontani dai valori, purtroppo misconosciuti o addirittura rinnegati, tipicamente europei. Già l'allargamento a Paesi di cultura e geografia, più banalmente, estremamente vicine all'Europa ha comunque determinato e sta determinando qualche problema proprio per l'eccessiva

è stato vissuto da sempre come il nemico storico delle nostre Nazioni, soprattutto di tutte le Nazioni europee che si affacciano sul Mediterraneo e non solo. Ricordiamo la visione presente nell'immaginario

i contrasti di una certa gravità tra l'Europa tradizionale e il Continente, cioè tutta la cultura e la storia della Turchia,

di queste popolazioni. Popolazioni che, come gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno tranquillamente dimostrato, sono ancora estremamente lontane dal pensare in un modo che sia solo lontanamente europeo. Basta vedere le manifestazioni degli ultimi mesi e l'atteggiamento che lo stesso Primo ministro turco ha nei confronti dell'Europa, quasi che l'Europa avesse un obbligo, non si capisce bene di che tipo, a far entrare la e se non la si fa entrare alle condizioni che hanno in mente quasi quasi sono loro che con un gesto di stizza si allontanano da noi. La Turchia, oltre a questa

completamente annientate. Ciò rappresenterebbe un inserimento che annacquerebbe o comunque farebbe diventare completamente diversa l'identità europea che tradizionalmente tutti noi abbiamo in mente. Certo, ci sono poteri forti che hanno tutto l'interesse a far entrare la Turchia in Europa; oltre a tutti i poteri economici che hanno fortemente investito in quel territorio e che comunque hanno in mente di gestire il mondo solo da un punto di vista economico, ci sono anche altre potenze politiche e militari; gli stessi Stati Uniti, nei confronti dei quali abbiamo un certo tipo di atteggiamento in altre situazioni, che non possiamo certo condividere per quanto riguarda la Turchia. Gli Stati Uniti sono a 12.000 chilometri dalla Turchia, la vedono esclusivamente come una base militare importante per gestire questa parte del mondo.

sociale ed economica del nostro Continente con l'inserimento di un entità così consistente, come l'entità turca, sicuramente avrebbe tutti questi tutti questi effetti, visti positivamente dall'altra parte dell'Atlantico. Noi però abitiamo qui ed è alla nostra realtà che dobbiamo pensare. Un'Europa con un'impronta prettamente economicistica, nella quale un euro forte riflette un'economia debole, contraddizione, questa, che sottolinea quanto sia stato inopportuno introdurre l'euro prima di aver raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, politica, sociale ed economica. Anche in questo caso viviamo quotidianamente dei paradossi economici che solo la politica

all'anno e che ha una moneta debolissima che ovviamente l'aiuta ulteriormente nella sua crescita economica; abbiamo gli Stati Uniti che comunque crescono al 4-5 per cento all'anno e che sono riusciti a diminuire imponendo la loro diminuzione del valore del dollaro rispetto all'euro. Abbiamo un'Europa che è un continente in via di deindustrializzazione, di invecchiamento della popolazione, senza grandi innovazioni tecnologiche, che cresce solo al due per cento all'anno e ha la moneta più forte del mondo: è evidente che c'è qualcosa che non quadra in questa Oltre tutto una moneta così forte, con un'economia così debole, in senso relativo ovviamente, rispetto agli altri Paesi del mondo, sta velocemente portando ad effetti ovvi: c'è un aumento delle importazioni, perché abbiamo una moneta forte, una diminuzione delle esportazioni, perché abbiamo una moneta forte, e tutto questo porta sostanzialmente ad una deindustrializzazione e comunque ad una riduzione della capacità economica complessiva del nostro Continente. Questo è spiegato solo dalla politica: mentre le altre potenze, parliamo della Cina e degli Stati Uniti, oltre ad essere potenze, hanno anche un'entità politica vera, e quindi la loro economia riescono a gestirsela direttamente, noi siamo, per così dire, terra di nessuno, un grande territorio puramente economico dove tutti fanno affari ma dove la politica, quella vera, che dovrebbe rappresentare gli interessi del popolo, non esiste. Il Trattato costituzionale, da tanto millantato come la soluzione alle gravi crisi di identità dell'Europa, per come è stato concepito può aggravare e non risolvere i problemi, e che le presidenze europee di turno vogliano continuare a mantenere quel documento sul tavolo negoziale appare come la peggiore scelta in questo momento. Se la presunta futura Costituzione europea è stata così pesantemente bocciata dai popoli che si sono potuti esprimere riguardo alla stessa (ricordiamo che dove non è stata bocciata è stata semplicemente perché non si è votato; infatti, sono convinto che se nella maggior parte delle Nazioni si votasse il risultato non sarebbe molto diverso da quello ottenuto in Francia e in Olanda), non è stato perché gli europei siano contrari all'Europa, ma probabilmente perché chi ha scritto quel tipo di Costituzione si è dimenticato di quello che gli europei normali pensano dell'Europa in cui vivono.

protestanti praticanti, ma significa semplicemente prendere atto di una realtà di fatto che è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo quello che siamo anche perché c'è stata questa storia nel nostro Continente, altrimenti saremmo stati un'altra cosa, e rinnegarlo, non metterlo volutamente nella Costituzione, è stato uno schiaffo che tutte le popolazioni che hanno potuto votare hanno fatto pagare bocciando la Costituzione stessa, per non parlare di altre cose che sono veramente contrarie al sentire comune. Nella bozza di Costituzione il matrimonio è indicato come un'unione di individui, senza specificare il numero e il genere. È evidente che ognuno ha i gusti che ha e ognuno fa quello che vuole nella vita, ma nel libro della legge, nelle tavole della legge non si possono non citare le cose normali, che fanno parte non della tradizione consolidata, per il gusto di dire che è un qualcosa che esiste da sempre, ma che è nella tradizione del buonsenso, del pensiero razionale tipicamente europeo. Avere indicato il matrimonio come unione di individui significa ovviamente - se ne sta parlando in queste settimane - aprire indistintamente al matrimonio tra persone dello stesso sesso, e devo dire a questo punto che sarebbe il minore dei mali. Infatti, un'autostrada, un'apertura enorme ad altre culture, tipo quelle che prevedono al proprio interno il matrimonio poligamico tra un uomo e più donne, perché a questo punto la Costituzione europea sarebbe già pronta ad accogliere questo tipo di organizzazione familiare. Manca, in definitiva, il coraggio, in questa Costituzione: manca l'orgoglio di essere europei. Questo è un libro della legge scritto non da chi è orgoglioso di essere di questi territori, ma da chi si sente un burocrate che deve regolamentare un qualche cosa da far approvare ai cittadini che sono ridotti a dei numeri, a delle tessere. Il mastodontico Trattato non garantisce più sicurezza: ricordiamo solo il mandato di cattura europeo, per cui noi che in Italia abbiamo già dei problemi con la nostra magistratura da domani potremmo essere arrestati a casa nostra perché abbiamo tenuto un atteggiamento da noi legittimo ma che è reato in un altro Paese europeo.

senatore Colombo ha una cultura a senso unico: quando parla lui, parla il vice Papa, quando parlano dalla sua parte tutti hanno la verità scolpita nella roccia; da questa parte ci sono solo gli analfabeti

*(FI)*. Basta! GALLI *(LNP)*. Non si può fare uno statuto, un codice civile e penale prima di aver omogeneizzato i comportamenti intellettuali, morali normali e quotidiani delle popolazioni. Non mette i produttori al riparo dallo strapotere e dai grandi interessi finanziari; non aumenta le garanzie sociali. Entrambe le questioni le abbiamo viste recentemente. Abbiamo assunto una posizione che magari i puristi del libero mercato possono non condividere, ma quando abbiamo parlato di dazi e quote ne parlavamo non perché pensavamo di poter fermare con delle leggi quello che è il normale andamento economico del mondo, ma porre delle regole significa come minimo frenare un eccesso di velocità di questo sviluppo: nessuno pensava di fermare la Cina o l'India

loro. In realtà, i politici europei non hanno mai difeso l'industria vera e popolare - mi sentirei di dire - delle nostre Nazioni e dei nostri Stati; hanno solo difeso la grande finanza e le grandi multinazionali.

una direttiva come la Bolkestein che avrebbe portato il *Far west* nelle nostre Nazioni. Si tratta di una direttiva per cui, se si vuole fare un *call center* in Italia, lo si poteva fare con le regole rumene a 200 euro al mese. A fronte di questa causa, la triplice sindacale non ha fatto neanche un minuto di sciopero. *(Applausi del senatore di protezione dei diritti civili e sindacali dei lavoratori. Sul discorso dell'energia abbiamo detto delle belle cose in questa Aula, però oggettivamente iniziative politiche europee vere non ne vedo.

molto poco. I cittadini europei non saranno messi nella condizione di capire di più, di potersi informare con facilità e si allontaneranno sempre più da questo leviatano incomprensibile e inutile. Il Trattato elaborato dalla Convenzione è intriso di relativismo etico e culturale; l'assenza di riferimenti a eredità culturali e religiose dell'Europa costituisce la formulazione giuridica dell'ideologia mondialistica che vuole gli uomini tutti uguali tra loro, senza tener conto della loro storia, delle loro tradizioni e del rapporto con il loro territorio. risultato che può essere anche condivisibile nella sua finalità ultima, ma deve tenere conto dei tempi degli uomini. Sicuramente tra 20, 30 o 50 generazioni il mondo sarà molto diverso da quello di oggi.

la cultura greca, il messaggio cristiano e la rivoluzione tecnico-scientifica. La prima ha introdotto la *forma* *mentis* teoretica, dalla quale sono derivate la filosofia e la scienza; ha inoltre elaborato il concetto di giusta misura, che è misurazione non aritmetica, ma fondata sui valori. Il messaggio cristiano ha portato significati prevalentemente morali e spirituali, ha elaborato il concetto di psiche, l'idea dell'uomo capace di intendere e di volere, l'importanza della cura dell'anima, il valore e la centralità dell'uomo come persona, in rapporto con gli altri e con Dio. Ha promosso i valori della tolleranza, dell'uguaglianza e della libertà, oltre che della grandezza dell'umile; ha messo al centro dell'esistenza umana il principio dell'amore. Oggi diamo tutto per scontato; ma, anche in culture peraltro avanzate da un punto di vista tecnico-scientifico, cose che noi diamo per scontate (la non divisione in classi, l'uguaglianza tra gli uomini, l'uguaglianza tra uomo e donna, come vediamo quotidianamente) non sono altrettanto presenti. La terza componente è la rivoluzione tecnico-scientifica, basata sul principio di verifica scientifica. Tali valori dovevano ispirare i legislatori europei, non solo astratti ideali politici e leggi economiche. Chi sostiene che l'Europa non debba avere una sua identità e debba invece aprirsi a tutte le differenze, senza porre alcun limite,

siamo estremamente orgogliosi di essere europei; vorremmo semplicemente un'Europa diversa. La sensazione è che molte delle persone che ci rappresentano a Bruxelles lavorino per altre forze, per altre potenze e non per gli interessi dell'Europa e degli europei.

Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, farò sfacciatamente un intervento molto strumentale. Lo dico io stessa, così non me lo rimprovererete poi. Ho scelto infatti di occuparmi dei problemi della parità tra uomo e donna, delle politiche di genere, che in Europa sono significative, tenaci e tuttavia rivelano ancora dei punti lontani dall'essere raggiunti.

parlamentari europee che non è male: Luisa Morgantini è vice presidente del Parlamento europeo, Angela Merkel presiede la Commissione e ci sono varie Ministre degli esteri. Sono molto orgogliosa che il nostro Paese abbia una Ministra per le politiche europee; tra l'altro, una Ministra amata e stimata. Pensiamo tuttavia di campare parassitariamente sulle glorie europee senza fare niente? È possibile mai che, dopo i peana sull'Europa, non ci sia nessuno che dica che, se facciamo una legge elettorale che non metta nelle sue priorità la necessità di avere strumenti efficaci (non prese in giro) per il riequilibrio della rappresentanza, facciamo pietà ai sassi e che tutte le cose che diciamo sull'Europa non hanno coerenza? Questa è una delle priorità: una legge elettorale che dica che non si può opprimere una minoranza (noi siamo addirittura la maggioranza dell'elettorato). Si può ragionare in questo modo? Fare inni alla razionalità come caratteristica della cultura europea e poi scordarsi repentinamente di tutto questo? Allora, io qui faccio un appello esplicito, forte, molto sentito al Parlamento, perché d'ora in avanti chiunque parli di legge elettorale non si scordi mai di dire che una delle sue priorità è il riequilibrio della rappresentanza, senza la quale tutto l'europeismo che si spreca a fiumi è una pura ipocrisia. Non possiamo continuare a campare parassitariamente sul fatto che in Europa le donne sono più presenti che nel nostro Paese. Non sono affatto orgogliosa di essere il fanalino di coda dell'Europa sotto questo profilo, assolutissimamente no! Chiedo con forza questa cosa e non la delego; non mi interessa che qualcuno (il Ministro o il Parlamento) scelga per me i modi della mia rappresentanza. Noi qui ci siamo e dobbiamo essere interpellate in modo trasversale e avremo delle indicazioni da dare su come costituire questa legge elettorale. Altrimenti, per l'appunto, si evidenzia una discontinuità logica e persino etica tra l'esibizione di buoni princìpi, di buoni sentimenti, di grandi ideali, persino di utopie straordinarie, e la miseria

perché dell'Europa questa è una delle grandi caratteristiche: si costituisce quando le donne sono tutte cittadine e avendo alle spalle l'esperienza dello Stato sociale, la forma più avanzata di Stato che si sia vista sul pianeta: uno Stato nel quale i diritti sociali sono universali, sono diritti comuni esigibili. È inutile parlare tanto di famiglia se poi non ci sono diritti esigibili;

che non può essere sostituito, per l'appunto, da interventi casuali, privatistici, non universali dove non sia previsto il diritto e la esigibilità del diritto stesso attraverso delle politiche.

e questo processo attraverso il quale vediamo formarsi un soggetto politico molteplice - perché l'anima dell'Europa è la molteplicità è la molteplicità - insegna come si fa a governare con la pace, che è il governo della molteplicità, non la sua riduzione, non la sua omogeneizzazione, non la sua repressione o una sua dimenticanza. Molteplicità di ordinamenti, dunque, di lingue, di culture, di religioni, che o convivono o diventano distruttive. Non ci ricordiamo più cosa sono state le guerre di religione in Europa? Una cosa terrificante. Cosa è stato, sotto il titolo di *Sacrum Imperium*, il conflitto per il potere politico? È possibile mai che non ci ricordiamo che l'Europa è stata il continente più insanguinato e più insanguinante, più cruento, che abbiamo portato dappertutto i nostri cosiddetti valori (la religione, le ricerche scientifiche, le scoperte geografiche) attraverso la violenza? Tutto questo ci si rivolta contro, ma nello stesso tempo diventa una straordinaria lezione. Se siamo in grado di dire che questo è un continente che si costituisce come soggetto politico attraverso la pace, la politica, la diplomazia, la trattativa, è un esempio straordinario per il mondo; attraverso lo Stato sociale, che è una forma dove il diritto è esigibile ed è diritto comune, e attraverso la presenza delle donne come cittadine, che per la prima volta si vedrà. Ho sentito qualcuno lamentare che i Padri in 18 mesi non sono riusciti a fare niente; succede che le donne in nove mesi fanno i bambini! Provate un po'. un po'. È meglio che ci siano anche delle madri, oltre ai padri, in Europa, perché i padri da soli pare che facciano poco, e qualche volta anche pasticci, per la verità. Voglio ricordare questo proprio per concludere che, se non abbiamo una sufficiente fantasia politica per capire che la conservazione, addirittura il culto della molteplicità, la capacità di affrontare le cose da molti punti di vista è la più straordinaria scoperta del pensiero politico contemporaneo ed è sicuramente uno dei grandi contributi del femminismo (perché quando si dice che i soggetti sono due, se sono due possono essere la serie infinita dei numeri, si deve rompere l'uno perché diventi possibile la molteplicità e non solo il pluralismo, che è la ripetizione dello stesso modello), se non riusciamo a mantenere questo, e per ciò bisogna che le donne siano un soggetto riconosciuto e non una *octroyée* di qualche dono o di qualche mazzo di mimose l'8 marzo (poi non se ne parla più fino all'anno successivo), credo che non arriveremo da nessuna parte: continueremo ad avere dei dei tentativi, delle speranze che si infrangono. Non volevo dire altro che questo. L'ho detto che era strumentale, ma mi pare sia una strumentalità con un qualche significato, almeno questa è la mia convinzione.

ci si innalza nell'uso del linguaggio ad una visione a 30.000 metri di quota dimenticando che proprio chi crede fortemente nell'Europa

con la caduta dell'ex Unione Sovietica, l'Unione Europea era sostanzialmente la seconda grande potenza mondiale: la Cina era ancora sullo sfondo e non era ancora entrata nella WTO; dell'India si parlava con curiosità;

con grande amarezza. Avremmo sperato, nella celebrazione del cinquantesimo anniversario, di dire qualcosa di diverso. Allora, con grande franchezza, proprio seguendo le indicazioni fornite dalla relazione, proviamo a parlare - ad esempio - di confini.

In fondo, stiamo ottenendo un risultato pessimo, vale a dire che la Turchia si allontana dall'Europa senza avere neanche noi il coraggio di rompere tale rapporto, magari dimenticando l'apportodato dalla Turchia alla NATO, ai sistemi difensivi, ilruolo geopolitico che quel Inoltre, signora Ministro,i Balcani sono il giardino di casa dell'Italia. Siamo molto preoccupati nell'osservare il disinteresse dell'Unione Europea verso i Balcani; siamo preoccupati nell'apprendere che tedeschi e inglesi lasceranno la Bosnia-Erzegovina e lasceranno la loro appartenenza alle truppe dell'Unione Europea. Sembra quasi che il Nord-Europa verso i Balcani abbia un atteggiamento critico dopo averci imposto alcune soluzioni: qualche volta bisognerà pur affermare che la crisi dell'ex Jugoslavia nasce da una certa non felice scelta della Repubblica federale tedesca in materia di riconoscimenti, peraltro assunta senza consultare l'Unione Europea. Abbiamo un problema come Italia: siamo i soggetti protagonisti e siamo ancora qui a disquisire con vecchi metodi e vecchi criteri. Mi perdoni, Ministro, so che lei crede nei tribunali penali internazionali - ci credo anch'io però è possibile che condizioniamo così pesantemente un rapporto con la Serbia, legato a fatti che certamente hanno un'incidenza nel giudicare la storia ma che sono di ostacolo allo sviluppo dei rapporti con la Serbia

che non si può separare oggi quello che è insito nella cultura serba, anche riconoscendo gli errori che, voglio dire, qualche volta bisogna riconoscere. Noi siamo andati in Kosovo con un grande compito che era quello di mantenere l'equilibrio tra le due comunità. Oggi questo non c'è. Oggi, a parte il nord del Kosovo, dove è abbarbicata una minima presenza serba, siamo lì a difendere le chiese ortodosse dall'aggressione dei musulmani e dell'Albania. c'è una responsabilità dell'Unione Europea, dell'Italia, della NATO, del multilateralismo che spesso questo Governo invoca. Anche qui, questo confine, questa parte dell'Europa deve entrare, ma in quale modo, con quali condizioni? Deve rappresentare un problema per l'Europa o deve rappresentare la grande occasione di sviluppo che sono state la Polonia, la Cecoslovacchia allora, e la Cechia e la Slovacchia oggi, o come sono ormai la Romania e la Bulgaria, ventiseiesimo e ventisettesimo Con quale spirito ragioniamo di allargamento dei confini? Ho un dubbio, che non è solo mio; viene da alcune osservazioni della politica britannica: stiamo forse costituendo un Commonwealth? Una comunità di popoli che si dà regole comuni per una convivenza certamente pacifica, socialmente evoluta in cui, economicamente, uno si sorregge all'altro, con una moneta unica che riesce ad aiutare anche Paesi che hanno difficoltà come noi ma che, al di là di questo sentire comune, non riesce a ritrovare in se stessa una capacità di essere anche forza politica, di essere forza militare? Non vale la pena (e qui vengo al Trattato costituzionale, perché sa, la riflessione ancora fino al 2008 - viva Dio! - non è certamente un grande successo; in fondo i *referendum* della Francia e dell'Olanda sono passati)

a trovare i responsabili? Questa è l'Europa che tutti insieme abbiamo costruito, sia chi vuole dare uno spirito, una missione quasi messianica alla costruzione dell'Europa sia chi, come noi, pensa con grande realismo alla costruzione di quello che anche noi da giovani sognavamo come un'occasione di grande riscatto di quest'Europa, fino ad avere un'Europa che di per sé, proprio perché è semplicemente, a mio giudizio, un Commonwealth*,* è incapace, per esempio a livello di *Doha Round*, di dare risposte. Ci chiedono cose, Ministro. Lei lo sa meglio di me che alcune cose le chiedono, anche di sacrificio all'Europa. Quando parliamo di aiuto ai Paesi in via di sviluppo, quando cerchiamo di investire o di fare investimenti per innescare processi di sviluppo virtuosi all'interno di Paesi poveri poi mettiamo le barriere sulle banane, sullo zucchero, sul cioccolato, cioè ci chiudiamo in una torre di avorio che difende gli interessi di un'Europa molto ricca e molto egoista in questo senso, allora siccome qui si è molto parlato di anima, anima è anche avere la forza di porsi come modello di comportamento, di mondo ricco, di mondo industriale, di mondo evoluto verso altre realtà che guardano certamente all'Europa con grande attenzione ma che non trovano in quest'Europa, molto legata a difendere i propri interessi, un discorso che sia aperto e diverso. Qui si è cercata l'anima. Non so definire né capire che cosa voleva Angela Merkel, ma mi domando, visto che c'è anche un'azione tesa a recuperare i giovani europei: come come si può immaginare di dare un'anima, una missione, un obiettivo, una forza capace di trascinare e di superare ostacoli in un'Europa che fa della filosofia della penitenza la sua filosofia? Possibile che quest'Europa sia colpevole di tutti i mali del mondo? Possibile che solo noi abbiamo distrutto il mondo, come se non avessimo dato al patrimonio dell'umanità la cultura nella storia europea, si sono conosciuti i genocidi più spaventosi, ma è anche vero che quest'Europa è uscita dalle sue tragedie senza nessuna cooperazione allo sviluppo di altri,

ha cercato strade diverse, si è inventata nuove politiche e nuove storie. Allora, perché continuare in questa filosofia della penitenza? Perché farci colpevoli di tutti i mali del mondo? Alla gioventù e alla gente alla gente che deve credere nel futuro come si fa a proporre una madre che ha tutte queste colpe? Avrà pure qualche virtù, qualche radice storica, culturale

nel Medio Oriente. Come si può affrontare un dialogo di civiltà quando *a priori* non si ha il coraggio di difendere la propria civiltà e la propria scala di valori? Perché un dialogo di civiltà è un dialogo fra due pari, che hanno radicato senso e scala di valori e che dialogano per trovare modelli di convivenza possibile, magari anche cercando di proporre modelli, come i nostri, che meglio di altri consentono la convivenza di differenze culturali, anzi le hanno profondamente esaltate.

di parlare seriamente di un *flop* terribile. Nel 2010 avremmo dovuto misurarci con questo grande mercato libero e comune. Non mi pare ci siano le premesse. Non c'è solo una responsabilità dell'Europa. Dobbiamo dirlo francamente: la sponda Nord dell'Africa ha certamente fatto grandi passi in avanti, ma da qui a quello che pensavamo in termini di libertà di mercato, di libertà di associazione politica o di pluralismo politico credo che ancora molta strada debba essere percorsa. Certamente nel processo di Barcellona la questione mediorientale e israeliana è un fatto che possiamo sforzarci di risolvere, ma non dipende da noi. Allora, perché continuare a sognare qualcosa che in realtà non è più uno strumento? E questi patti che noi facciamo come Europa

La risposta del Governo italiano, così filoeuropeo, è stata lo spacchettamento di una serie di deleghe ministeriali, per cui è difficile immaginare la Strategia di Lisbona sul Governo italiano, perché competenze così difformi certamente non aiutano il processo europeo. Andando ancora oltre, si affronta il problema dell'energia; la Germania l'ha posto, ma tutti noi sappiamo come l'interpretazione del libero mercato in Francia e in Germania sia profondamente diversa rispetto

una forte coscienza di sé, della propria identità nazionale, della propria capacità di operare all'interno dell'Europa. Noi ci auguriamo che chiunque succederà a Jacques Chirac e a Dominique de Villepin affronti in maniera diversa il rapporto con l'Europa. però, è inutile parlare di complesse politiche di sviluppo sull'energia e sulle grandi infrastrutture fino a quando sopravvivono sistemi così profondamente diversi, che in molti casi impediscono,

non è un fatto di cronaca, ma appartiene ai grandi mutamenti che stanno avvenendo nel ventunesimo secolo. Come può l'Europa rispondere solo con la polizia, faticosamente, con fondi assolutamente ridicoli e assurdi rispetto agli impegni, e scaricando su Spagna e Italia la responsabilità di gestire fenomeni riguardanti continenti di 800 milioni di persone? Come può l'Europa ragionare in questo senso, lasciando aperte le strade, praticamente, a questi fenomeni, non controllandoli, non avendo nemmeno la forza, l'intelligenza o la capacità di misurare le esperienze britanniche e francesi?

Vogliamo parlare del motivo per cui l'Europa non riesce ad organizzare una sua autonoma capacità di difesa, se non all'interno di un sistema NATO? Tale sistema, ovviamente, è ben diverso da un sistema di capacità di autodifesa anche per la presenza di di un *partner* invadente, importante, pesante e spesso lontano dalla nostra cultura e dal nostro modo di porre i problemi.

della NATO e dell'Unione Europea impegnano politicamente l'Europa a risolvere un problema di frammentazione di uno Stato e di creazione di Stati - perché non dirlo? - criminali (e sappiamo perfettamente quali siano questi

sulle capacità di difesa dell'Europa o immaginare situazioni oggi difficili da immaginare, perché l'Europa non si fa carico almeno della situazione dei Balcani?

Il Cancelliere tedesco, in qualità di presidente di turno dell'Unione, ha preannunciato che si farà direttamente carico di riassumere le posizioni dei diversi Stati europei in un unico documento, nel quale saranno sottolineati i successi dell'Europa e sarà indicata la volontà di superare l'attuale *impasse* istituzionale prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2009. L'Italia ha aderito a questa posizione. Il vero problema, tuttavia, non è quello di arrivare al 25 marzo, ma di scegliere la direzione verso cui condurre l'Europa in vista dell'appuntamento del 2009. Essendo ben chiaro a tutti che abbiamo di fronte due anni cruciali nei quali l'Europa dovrà trasformarsi se vorrà sopravvivere. Cominciando col risolvere la principale aporia di fondo che la contraddistingue, il fatto cioè che, come ricorda Garton Ash, «l'Europa è un grande catalizzatore di democrazia, ma lei stessa non è molto democratica». E in effetti la costruzione del nuovo Trattato europeo è caduta proprio in due *referendum* popolari; a seguito dei quali si è aperta una fase pudicamente definita di moratoria, che i principali attori della scena europea sembrano incapaci di superare. Molti hanno avanzate ricette, ma nessuna sembra quella risolutiva: terminare il ciclo delle ratifiche di un Trattato che è già stato respinto sarebbe insensato; scrivere un nuovo Trattato potrebbe esporre al medesimo fallimento; condensare in pochi fondamentali punti il terreno di una scelta comune, una sorta di minitrattato, come sostiene Nicolas Sarkozy, potrebbe essere forse la via d'uscita più realistica.

che, ancor di più dopo l'allargamento, non dispongono della capacità decisionale adeguata alle sfide che devono fronteggiare. Basti solo pensare ai tempi di reazione in caso di crisi o alla tripartizione dei poteri (Consiglio, Commissione e Parlamento), che conduce più a un sistema di rivendicazione di competenze che a un centro di decisione unitario e riconoscibile. Senza trascurare il fatto che il comune cittadino europeo, proprio a causa di tale complessità, non è in grado di descrivere le istituzioni europee né di identificare il titolare di un potere sovrano (ammesso che un potere sovrano esista). Su tutto ciò il nostro Governo tace. Ma essere europeisti non significa adottare la politica dello struzzo e far finta che vada tutto bene o andare a rimorchio delle scelte altrui. Se si vuole bene all'Europa, occorre essere impietosi nella diagnosi dei suoi mali e lungimiranti nella terapia; e smettere di essere autoreferenti e considerare i mali d'Europa come se non fossimo europei: vista dall'esterno l'Europa funziona e, soprattutto, giustifica sua esistenza? Basti considerare i due fronti principali della crisi: la politica estera e di difesa e la politica monetaria. In politica estera ogni Stato è geloso della propria sovranità e l'Europa è un nano nello scenario mondiale: la memoria va alla vicenda dell'ex Jugoslavia, un genocidio nel cortile di casa. Quanto alla politica monetaria, la mancanza di un potere sovrano fa sì che l'euro sia una valuta senza uno Stato, dato che, come ricorda Benjamin Cohen, «anche se i membri dell'unione monetaria hanno una politica unica non hanno interessi unitari» poiché, a differenza dei banchieri centrali, il *board* di direzione della BCE, a causa della sua composizione rappresentativa dei singoli Paesi membri, «non va verso il razionale di una politica monetaria integrata, ma tende a rinazionalizzare la politica monetaria europea», dato che i suoi componenti, oltre al fatto di essere troppi e quindi di evidenziare la circostanza drammatica che manca un «*Mister* euro», un centro cioè di decisione unica in caso di crisi (in caso di crisi valutaria occorrerebbero giorni per mettere d'accordo tutti e per reagire), più che rappresentare interessi comuni, sono portatori di specifiche attenzioni verso i singoli Stati. E la questione - inutile nasconderlo - è resa più grave dall'allargamento. Il tutto perché l'Unione contiene in sé due aporie logiche, che occorre risolvere se si vuole arrivare a una revisione del Trattato che abbia una qualche possibilità di successo: l'allargamento in mancanza di una *governance* adeguata a conciliare i contrapposti - e spesso egoistici - interessi nazionali e a fronteggiare le situazioni di crisi, in mancanza di un centro unitario di *crisis management*, e, in campo economico, la contraddizione tra i mezzi e i fini, costituiti i primi dalla politica monetaria della BCE e dall'attività regolatoria dell'Unione e i secondi dall'obiettivo di politica economica dello sviluppo dell'area comune. Su quest'ultimo tema sarà opportuno soffermarsi, anche in considerazione del fatto che, in mancanza di un presidente o di un altro simbolo visibile, la moneta ha finito per assumere il valore di unico simbolo dell'Europa. Ma la moneta da sola non può essere l'Europa. Non è l'interesse superiore per il quale soffrire e combattere. La moneta è uno strumento. Non è un fine. È anche uno strumento insidioso: i cittadini possono anche non rendersi ben conto di una crisi politica in corso, ma ognuno si accorge subito ed è direttamente coinvolto in caso di crisi economica. L'Unione Europea, oggi, si è affidata interamente per il proprio funzionamento e per la propria visibilità ideale alla moneta, per tal via rischiando di condizionare il suo successo esterno a dinamiche interne. Ma non si può caricare di valore uno strumento che nasce su un equivoco di fondo. Anzi, su un duplice ordine di equivoci: da una parte, l'euro è un potente strumento per aprire i mercati, ma gli Stati europei temono i mercati aperti; dall'altra, l'Europa ha bisogno assoluto di sviluppo per garantire agli europei almeno il mantenimento del loro attuale tenore di vita nell'era della competizione globale, mentre la moneta comune funziona come strumento per frenare la crescita, poiché l'obiettivo della BCE è quello di tenerne alto il valore. Anche perché l'Euro è nato con grandi ambizioni esterne, ma ha finito per essere relegato al campo degli strumenti di politica interna. Per il premio Nobel Mundell, l'euro avrebbe cambiato i rapporti di forza tra le monete, e probabilmente uno degli obiettivi iniziali era proprio quello di contrapporre l'euro al dollaro. Ma in questo modo si rischia di valutare il successo o l'insuccesso dell'euro esclusivamente in funzione dello stato di salute o di crisi del dollaro. Se è così, tuttavia, la grande ambizione globale della nostra moneta risulta frustrata dal suo tuttora scarso ruolo internazionale. A cinque anni dalla sua entrata in vigore l'euro non ha ancora, come ricorda sempre Cohen, acquisito quel prestigio interno ed esterno che deriva dall'indiscussa e diffusa percezione del godimento di tre attributi: la stabilità dei fondamentali dell'economia sottostante, la convenienza ad utilizzarla come strumento delle transazioni e la generale accettazione come strumento di pagamento. Quanto alla stabilità, come ricorda Anna Schwartz, «le prospettive dell'euro sono sotto le nubi di un immenso sforzo finanziario che i governi dovranno sopportare nei prossimi 50 anni, se vorranno onorare la loro promessa di pagare pensioni generose e le spese sanitarie di una popolazione che invecchia», poiché ancora non è dato sapere se «i paesi dell'EMU sceglieranno la via delle riforme tempestive o abbandoneranno la disciplina monetaria per far ricorso all'offerta di denaro per finanziare la spesa». Non solo. In Europa non si è neppure in presenza di un solo modello economico-sociale, come lamenta Erik Jones, ma addirittura di quattro, secondo il calcolo di André Sapir. Ogni zona, se non ogni Stato, dispone di un suo modello e lo difende. La realtà è che «l'EMU attualmente non rappresenta una unione di uguali». Come dimostra con evidenza il fatto che il Patto di stabilità e crescita contiene al suo interno una vera e propria bomba ad orologeria. Da una parte, definisce una regola generale di convivenza, tal che la sorte di ogni Paese è inscindibilmente legata al buon comportamento di ciascuno degli altri, rispetto al quale ogni singolo *partner* europeo ha però interessi spesso divergenti. Dall'altra, affida ad un mero meccanismo di *governance* finanziaria - la regola astratta (c'è chi la definì stupida) del 3 per cento, che non differenzia il livello di entrate e di spese, né tra spese buone e spese cattive - lo strumento per valutare la coerenza delle scelte economiche rispetto agli obiettivi generali, che, a questo punto, non esistono più, essendosi i mezzi sostituiti ai fini. È un tema che evidenzia una contraddizione di fondo insita nella scelta dell'unificazione europea per via monetaria: quella di aver privilegiato i meccanismi istituzionali rispetto all'efficienza del sistema. L'aver perso l'occasione, come ricorda James Buchanan, per realizzare ciò che Hayek definiva «un regime di moneta competitiva», e che avrebbe comportato effetti meno drammatici per il pubblico e «non avrebbe consentito decisioni discrezionali da parte di autorità esistenti solo sulla carta». Ma è proprio questa la scriminante tra ciò che sta dietro il dollaro e ciò che blocca la riuscita dell'euro. Come precisa Hans Martens, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, una quota variabile tra il 40 e il 55 per cento del PIL europeo è speso in azioni collettive.

quando non anche all'adozione di specifiche regolamentazioni disincentivanti da parte di singoli Paesi. E d'altronde, il fatto che il più importante mercato finanziario europeo sia quello britannico, cioè di un Paese che non appartiene all'area euro, la dice lunga sull'argomento. D'altra parte, la funzione della BCE in questi anni è stata quella di mirare al rafforzamento della moneta, tenendo sotto controllo l'inflazione; il che significa una politica monetaria restrittiva e di tassi relativamente elevati (vedi l'ultimo rialzo al 3,75 per cento e, dunque, una limitazione delle possibilità di sviluppo economico. La stabilità ha prevalso sullo sviluppo; e, se certamente è difficile che la moneta comune possa avere successo senza un'adeguata crescita della domanda interna, non vi è dubbio che all'euro sia mancato in questi anni il sostegno popolare, non solo per gli effetti del *change over* sui portafogli delle famiglie, ma soprattutto perché non vi è stata un'adeguata informazione da parte dei politici europei; cosa in realtà che non si poteva pretendere, dacché essi avevano delegato ad un organismo tecnico un loro potere sovrano. In sostanza, un processo tutto interno. «Il problema di lungo termine per la BCE è che l'Unione monetaria era qualcosa che l'*élite* politica di Francia e Germania ha ricercato. Ma non un cambiamento desiderato dagli elettori»: così ancora Schwartz. Circa, infine, la questione dell'accettazione, occorre essere assai cauti. Infatti, l'attuale forza dell'euro - dopo un primo periodo di oscillazione - «è spiegata dal fatto che gli investitori europei hanno sostituito l'euro al dollaro nella composizione del loro portafogli», ma la conseguenza sarà che, «se va così, arriveranno più esportazioni asiatiche, i risparmi europei resteranno a casa e i guadagni sui risparmi declineranno e così la crescita dell'economia europea si indebolirà»,(ho citato nuovamente Schwartz). Senza trascurare il fatto che un euro forte crea problemi alle nostre esportazioni. Ma è un euro forte solo nominalmente, dato che non riflette le vere condizioni dell'economia europea: basti badare al fatto che, a dati 2005, venivano regolate in euro il 37 per cento delle transazioni mondiali, una percentuale certo superiore rispetto a quella della principale moneta europea prima dell'unificazione, il marco tedesco, che si attestava al 30 per cento, ma decisamente inferiore rispetto al 53 per cento rappresentato dalle monete dei Paesi che ora appartengono all'area euro. E il dollaro resta forte, dato che è regolato in dollari il 50 per cento dell'*export* mondiale, il che rappresenta circa il doppio della partecipazione americana all'*export*. Quindi, a livello mondiale l'euro è sottodimensionato rispetto al suo potenziale. D'altra parte, al momento dell'adozione dell'euro non si assunse con chiarezza una decisione circa il fatto che la nuova moneta si dovesse porre in termini di competizione oppure di collaborazione rispetto al dollaro. La sua gestione concreta la sta orientando ad essere uno strumento di pagamenti competitivo, ma la realtà dei mercati dimostra che essa non è in grado di vincere una sfida tanto ambiziosa. E non lo è perché il sistema economico prevalentemente diffuso negli Stati europei non è in grado, al momento attuale, a causa delle contraddizioni già dette, di offrire una stabile prospettiva di duraturo successo nella competizione globale (basti considerare le proiezioni sull'andamento del PIL e del PIL *pro capite* da qui al 2050). E poi, cosa accadrebbe se gli avanzi della bilancia dei pagamenti cinese si riversassero in investimenti in titoli europei? Siamo attrezzati per rischiare un deficit di livello paragonabile a quello americano attuale senza disgregare l'Unione? Meglio dunque adottare finalmente una decisione razionale e abbandonare il modello di un euro come moneta competitiva rispetto al dollaro e concentrare gli interventi su quanto è necessario per rendere l'euro una moneta accettata dai cittadini europei. A cominciare dalla costruzione di un legame tra moneta ed economia reale. Siamo tutti convinti che l'euro rappresenti un processo irreversibile, una realtà rispetto alla quale non esiste neppure un meccanismo di uscita e che quindi va accettata. Ma va governata. E se ciò che esiste è l'euro, da esso dobbiamo partire, adattando la *governance* della nostra economia e delle nostre istituzioni alle conseguenze logiche che comporta l'adozione - e, se vogliamo, la sfida - di una nuova moneta. Per muoversi lungo questa direzione occorre intraprendere un'azione che mira a cogliere quattro obiettivi. Innanzitutto, per sanare la contraddizione tra stabilità e sviluppo, è preliminare orientare il sistema economico europeo, e con esso le economie nazionali, allo sviluppo. E, come abbiamo visto, per andare in questa direzione è necessario rimuovere la spada di Damocle che pende sulla testa degli europei e che consiste nell'attuale incapacità di molti Governi del vecchio continente di realizzare quelle indispensabili riforme strutturali, a cominciare da pensioni e sanità, che pregiudicano la reale possibilità di fare dell'euro una moneta competitiva e attraente sui mercati internazionali. Anche i Paesi che da ultimi si sono mossi su questo fronte hanno adottato soluzioni tutto sommato deludenti: la Germania ha elevato sì l'età pensionabile a 67 anni, ma il nuovo regime sarà pienamente in vigore solo nel 2020. Se questa è la realtà, occorrerebbe porsi il problema di una nuova interpretazione del principio di sussidiarietà, una volta che ci si è resi conto che i singoli Stati non sono da soli in grado di realizzare riforme che sono indispensabili per il benessere collettivo. Non c'è alcun motivo per il quale a livello europeo si decidono i comportamenti di finanza pubblica di ciascuno Stato e si rinuncia invece a porre le linea guida dei fondamentali economici sui quali si basa la finanza pubblica. Se il 3 per cento vale per tutti, valga per tutti anche una medesima età pensionabile. In secondo luogo, una volta riconosciuta la «stupidità» del patto di stabilità e crescita, se ne traggano le conseguenze. Si passi ad un patto ragionato, nel quale non vengano trattate in modo uguale situazioni diverse e nel quale non sia evidente che le sanzioni vengono inflitte ai piccoli e interpretate per i grandi. E siccome il 3 per cento non ha lo stesso valore economico indipendentemente dal livello di pressione fiscale e di spesa pubblica, si passi ad un sistema nel quale l'obiettivo europeo riguardi il livello complessivo della spesa e l'onere totale delle imposte. Magari consentendo a ciascun cittadino europeo di scegliersi il regime fiscale preferito nell'ambito di quelli disponibili nel panorama europeo. Dalla competizione tra sistemi nascerebbe anche la competitività del sistema europeo nel suo complesso. Ciò presuppone, ovviamente, che non vi debba essere una *governance* europea delle tasse, ma solo delle regole, a cominciare (ed è questo il terzo punto) dalla prefissione di un meccanismo di regole omogenee per i mercati finanziari. Sono a tutti note le ragioni per le quali una *Antitrust* europea rischierebbe di non funzionare in modo efficiente e capillare e per le quali sono state mantenute le Banche centrali dei singoli Paesi, ma occorre interrogarsi se questo schema non finisca per agevolare la difesa degli interessi nazionali - a volte egoismi - piuttosto che salvaguardare quello prevalente della libera circolazione di persone e di capitali. Da ultimo, è indispensabile snellire la *governance* della BCE, rendendola organismo non più rappresentativo degli interessi nazionali, ma adeguato a intervenire tempestivamente in caso di crisi. Risolvendo con l'occasione la questione se la Banca possa o meno funzionare come prestatore di ultima istanza. Ma la struttura della BCE non è tutto. Senza una modifica dei meccanismi istituzionali dell'Unione si potrà fare ben poca strada. Un sistema di comando che prevede la contemporanea esistenza di tre organi contrapposti - Consiglio, Commissione e Parlamento e un sistema di decisione sostanzialmente unanimistico, più che agevolare le decisioni, sembra preordinato a incentivare l'immobilismo. Oltre che incomprensibile sotto il profilo della logica, forse questo meccanismo poteva funzionare nell'Europa dei fondatori, ma in un'Unione a 27 costituisce un vero e proprio pericolo. Se l'Europa non sarà in grado di decidere autorevolmente e rapidamente, sarà costretta ad andare al traino della parte del mondo che si muove e, col tempo, perderà anche quella sua peculiare caratteristica di faro della civiltà che fino ad oggi l'ha contraddistinta. Per ottenere questo risultato occorre che ciascuno rinunci a qualche rendita di posizione e che finalmente la politica si riprenda un ruolo a cui da troppo tempo ha abdicato. La politica deve semplificare la politica europea. Come direbbe Altiero Spinelli, dalla Babele si deve tornare all'Europa dei padri fondatori». È tempo, signor Presidente, di abbandonare lo schema dell'Europa dei Governi e tornare a quello dell'Europa dei popoli.

Signor Presidente, signor Ministro, credo che la scheletrica risoluzione della 14a Commissione,

e denso di argomenti (taluni di essi meritano una rilettura sul testo scritto), un dibattito che conclude anche per il nostro Senato una pausa di riflessione: quella pausa di riflessione che fu decisa dopo le sconfitte referendarie di Francia e Olanda; sconfitte che non hanno riguardato solo quei Paesi e quei Parlamenti ma tutta l'Unione Europea e tutta la sua intera storia che cominciò nella primavera di 50 anni fa. Una pausa, perciò, tutta interiore, un dovere di ripensare come siamo, da dove abbiamo cominciato, dove andiamo; tutta interiore perché l'ingranaggio ha continuato a funzionare, perché la spinta integrazionistica, messa in moto mezzo secolo fa, ha continuato ad andare avanti con la sua logica. Basta leggere le impegnative conclusioni del Consiglio europeo di pochi giorni fa, l'8-9 marzo, per capire che le difficoltà della crisi non hanno travolto la missione, che è quella di guardare non solo dentro al nostro continente, ma dal nostro continente al mondo intero, una Regione multistatale che usa la forza di persuasione che le proviene dai suoi 500 milioni di cittadini, ma questa volta per assumere un ruolo guida nella protezione internazionale del clima. Questa visione, queste ambizioni, questi programmi, non sono certo quelli di un organismo in letargo. Al contrario, l'Unione Europea cerca per la salvezza fisica del pianeta (viene in mente il «*De rerum natura*» di Lucrezio Caro) un ruolo guida; e lo trova, quali che siano le difficoltà del suo ordinamento interno. Lo trova nella crisi climatica, così come nelle altre operazioni sotto il segno multiforme della sicurezza in cui è impegnata; da un lato, la missione di interposizione che sta consentendo una tregua, difficile e fragile, certo, ma una tregua, in Libano; dall'altro lato, la missione di cooperazione giudiziaria, di polizia, di contenimento dell'immigrazione clandestina, missione che si sta sviluppando a livelli normativi ed operativi in tutta l'area dell'Unione. E tuttavia, malgrado questo movimento continuo sui punti così sensibili della sicurezza ambientale, energetica e politica, abbiamo avvertito un dovere di riflessione per ripensare le basi, le fondamenta istituzionali che consentono questa azione, questo «eppur si muove». E noi capiamo che questo andare avanti e questa crisi hanno paradossalmente la stessa radice, sono causati l'uno e l'altra da una incompiuta sovranazionalità. Ecco, la pausa di riflessione ci ha consentito di vedere meglio nel problema della sovranazionalità e di capire che la forza giuridica della sovranazionalità si ritrova tutta intatta anche negli accordi intergovernativi nel quadro comunitario. Vi è tutta una pazienza europea da esercitare perché vi sia l'evangelica maturazione dei tempi per procedure giuridiche che si azionino con il meccanismo democratico della maggioranza. La democrazia della sovrastatualità i suoi ritmi e la sua progressione giuridica; non sopporta strappi, perché le istituzioni europee hanno solo 50 anni e le istituzioni statali ne hanno 500. Certo, di fronte alla ratifica di 18 Stati su 27, raggiunti i due terzi che nella comune civiltà giuridica europea consentirebbero di approvare qualunque Costituzione statale, vi è una impazienza di procedere di procedere al completamento di quell'ordinamento costituzionale che già formalmente e materialmente esiste in Europa. Esiste dal 1957, quando noi europei abbiamo deciso che certe leggi non le fanno più i Parlamenti nazionali ma le istituzioni normative comunitarie; quando abbiamo deciso che la Corte di giustizia interpreta il dritto per tutti i cittadini europei; da quando, cioè, abbiamo deciso che sono cambiate le nostre Costituzioni, perché le Costituzioni possono cambiare solo per effetto di fenomeni di natura costituzionale. E dobbiamo aggiungere che il fenomeno comunitario ha cambiato anche la conformazione interna degli Stati. La politica di coesione dell'Unione ha guardato più in là degli Stati Nazione, ha chiesto interlocutori territoriali a cui affidare gli interventi di area. 50 anni fa solo la Germania tra i sei fondatori aveva un assetto federale; oggi il regionalismo, con spinte accentuate verso il federalismo, è caratteristica comune degli Stati europei, sotto la spinta dell'Unione. Ma nel procedere per cumuli e stratificazioni, per successivi trattati, l'ordinamento costituzionale ha bisogno di una revisione profonda dei suoi meccanismi. Le ragioni del Trattato di Roma del 2004 restano perciò intatte. La pausa di riflessione ci ha permesso semmai di scarnificarle e di individuare quelle veramente essenziali. È il compito che si è data la cancelliera Angela Merkel; un compito che è nostro dovere non turbare. Dobbiamo fare attenzione a non contribuire anche noi ad aprire intempestivamente il vaso di Pandora delle rivendicazioni, come ci ha ammonito il nostro Presidente della Repubblica. Dobbiamo essere anche pronti a fare valere, se una seria apertura di negoziato vi sarà, le nostre posizioni nazionali e fra queste posizioni, di fronte ad eventuali muri e steccati di altri, vi potrebbe essere anche l'opzione dell'Europa della diversità, quella cioè d'organizzare, dentro il quadro istituzionale comune (Parlamento, Consiglio, Corte di giustizia, Commissione), forme di più intensa cooperazione tra gli Stati che vogliono andare più in fretta nell'integrazione istituzionale e nei risultati, come è stato per l'euro e come è stato per l'abolizione dei controlli di frontiera interna. La democrazia della sovranazionalità è anche nella capacità di far valere i diritti di una minoranza di Stati o di una maggioranza impedita dall'ostruzionismo di minoranza a sfruttare tutte le possibilità dell'integrazione, ferma la fedeltà all'impresa comune. Nasce da qui anche l'urgenza del provvedere, prima della scadenza democratica delle elezioni europee del 2009. Ma la democrazia della cittadinanza sovranazionale sarebbe un guscio vuoto se essa non fosse nutrita di contenuti ed evidenze che mordano, per così dire, lo stesso modo di vivere degli europei. Vi è oggi in Europa la rimessa in causa di un modello storicamente glorioso che è stato ed ancora è il modello sociale europeo. Sappiamo, anche troppo, come esso venga messo in discussione per la sua sostenibilità. Quello della sostenibilità è un problema serio che discende dall'organizzazione interna e internazionale del lavoro, da condizioni, ritmi e durata di vita lavorativa e da questioni demografiche assai importanti. E tuttavia, accanto al problema della sostenibilità, vi è un grande problema di ammodernamento del modello sociale europeo. Quando, dopo la Dichiarazione di Berlino del 25 marzo, si aprirà una fase negoziale, nei termini in cui si aprirà, sarà bene che il nostro Governo tenga conto

di cui parla Carlo Azeglio Ciampi, dell'armonizzazione contro il *dumping* fiscale, di tutele contro il *dumping* sociale, di una normativa quadro per i servizi di interesse generale. Ne abbiamo di recente constatato la necessità, parlando nella nostra Commissione dell'eventuale liberalizzazione dell'ultimo miglio del servizio postale. Ma, se Delors può sembrare - e non lo è un profeta disarmato, certo non può essere considerato tale Jean-Claude Juncker, nella sua posizione di Presidente dell'Eurogruppo, cioè del gruppo dei Ministri dell'economia dei Paesi dell'euro. Ebbene, Juncker, con la e il tempismo che gli sono propri, ha posto sul tappeto europeo la grande questione della redistribuzione dei frutti della crescita, senza rimettere in causa il principio di un'evoluzione salariale in linea con la produttività. Il Presidente dell'Eurogruppo ha però posto il problema dell'adeguamento dell'esame degli effetti della ripartizione tra utili e salari a livello macroeconomico. Se riusciremo ancora a organizzare un dibattito come questo, noi chiederemo che accanto al Ministro per le politiche comunitarie sia chiamato a rispondere il Ministro dell'economia. L'attuale titolare si confronta oggi con il grande tema della crescita economica, con l'esperienza di chi ha vissuto le preoccupazioni e le misure della stabilità monetaria. Signor Presidente, la nostra risoluzione impegna anche il Governo ad una riaffermazione dei valori che devono guidare il processo di Unione Europea. Tragiche e recenti esperienze ci devono insegnare che non vi può essere democrazia politica senza che, nello stesso tempo, sia introdotta una democrazia della cittadinanza. Non ci può essere separatezza fra modello di democrazia e sistema dei valori e dei diritti. Quello che dobbiamo difendere nell'Unione è un modello di democrazia integrata; una democrazia in cui ogni istituto, ogni procedura democratica sia legittimata da un'effettiva sfera correlativa di diritti e doveri soggettivi o collettivi ed in cui, viceversa, l'effettività di ogni diritto sia assicurata attraverso meccanismi democratici attivati dal basso e non sulla mera base di enunciazioni ottriate.

si voglia alludere, cioè al fatto che la sovranità democratica non può essere separata dalla sovranità dei diritti, dalla loro reciproca fertilizzazione, e che l'esportazione della democrazia non può essere concepita senza tener conto del territorio vitale e valoriale sottostante. Non a caso, nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, firmata a Nizza nel dicembre del 2000, si dice che l'istituzione della cittadinanza europea è possibile solo in quanto l'Unione l'Unione ponga la persona al centro della sua azione; la persona come alfa e omega della nostra civiltà europea, il nodo attraverso cui passano - sono ancora parole del Trattato - «le eredità culturali, religiose e umanistiche» della nostra storia. Sono le parole del Trattato del 2004, che ha anche una non retorica grandezza quando indica nell'Europa lo spazio privilegiato della speranza umana.

ci permettiamo di ricordare questa virtù al nostro Governo nell'antica certezza che la speranza, alla fine, non ci deluderà.

contrario, anzi c'è la consapevolezza della grandezza dell'eredità religiosa cristiana. Non vi è dubbio, questo è del tutto evidente. Non ci possiamo nascondere dietro una storia che vede nella questione cattolica, nella questione religiosa, un elemento di confronto continuo e positivo.

lavorare sulla nostra identità. Ma l'identità dell'Europa deve essere l'identità di una grande capacità, come dice la Merkel, di mettere insieme le diversità, la tolleranza. Forse vi è bisogno di più della tolleranza, una

sul *referendum* consultivo da abbinare alle elezioni europee. Credo si tratti di uno strumento di lavoro su cui impegnarsi e riflettere seriamente. Ho sentito però anche la capacità di combinare combinare questo senso di Europa ad un richiamo a restare con i piedi per terra. Noi siamo un Paese molto europeista - qui lo abbiamo detto tutti - però, colleghi, la mia frustrazione, che immagino sia anche la vostra,

i motivi fondatori di 50 anni fa sono rimasti esattamente gli stessi, ovviamente adeguati alle esigenze del 2007. I nostri padri e le nostre madri fondatori hanno pensato, nell'idea della comunità, ad un qualcosa che sapesse evitare le guerre tra di noi, che sapesse costruire un soggetto politico basato sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulla persona nei suoi diritti e nei suoi doveri al centro di una costruzione, e che sapesse produrre sviluppo. A me pare oggi di poter constatare che tutti questi tre cardini rimangono, ma aggiornati al 2007; oggi il problema non è più probabilmente quello di guerre tra di noi, perché abbiamo messo in moto sistemi tali che forse non sono neanche più pensabili, ma ci sono ci sono molto vicino, in Regioni che aspettano dall'Europa e da noi qualcosa che finora non siamo stati in grado di dare: una politica estera comune, una maggiore presenza sullo scenario internazionale. Se penso alla democrazia,

abbiamo esercitato (forse male, a volte, forse un po' troppo burocraticamente), questa attrazione ad un sistema di democrazia e di regole sia una delle politiche più positive: l'allargamento - ben venga se riusciremo poi a portarlo a termine - - ha fatto guardare all'Europa milioni di persone che uscivano obiettivamente da una situazione di non democrazia e di oppressione. Se poi penso allo sviluppo economico, credo che rimanga il terzo pilastro. Oggi, però, sviluppo economico vuol dire anche e soprattutto una proiezione globale, vuol dire soprattutto una posizione europea

ci siamo messi insieme e siamo diventati 27 membri sono gli stessi ma vanno adattati al mondo che è cambiato e che chiede un maggiore protagonismo della politica europea e dell'Europa: non l'Europa delle Patrie e delle Nazioni, ma l'Europa degli europei.

o a Strasburgo; ci va volentieri, ma non è questo il punto. Ho sempre pensato che la nostra delegazione a Strasburgo sia la terza Camera e dovremmo trattarla in questo modo.

perché sa adattarsi; a volte sa anticipare i tempi, altre sa perlomeno adeguarsi. Questa è la forza che ha portato altri ad essere attratti, a non vedere mai porte chiuse.

con molti Paesi, ad esempio del Sud del Mediterraneo. Credo che occorra ribadire che l'Europa sia un processo, che la nostra identità sia la democrazia

che sono poi quelle che fanno sì che si passi da una visione al modo vero di poter vivere insieme. Con questo spirito, voglio ringraziare ancora tutti coloro che sono intervenuti, anche quelli più critici che hanno dato comunque suggerimenti importanti: ad esempio,

risposta. Essa riguarda una situazione abbastanza preoccupante nel Comune di Tiriolo, dove si sono verificati frane e smottamenti che mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini di quell'abitato. Essendo trascorsi diversi mesi, sarebbe opportuno che i Ministri interessati ci dessero una risposta.